che è capitato nelle ultime ore: il Senato accademico dell'Università di Torino ha deciso di dire no ai progetti di cooperazione con Israele,

elementi preoccupanti del mondo accademico, come la lettera dei 1.400 accademici che chiedevano alle università, proprio su questo tema, di prendere una posizione; sostanzialmente, un vero e proprio boicottaggio accademico.

comportamento quasi al limite, che potrebbe essere considerato figlio di quell'ondata di antisemitismo che purtroppo abbiamo visto arrivare in Europa ed essere sempre più forte, dimenticando che le collaborazioni scientifiche e gli scambi tra gli studenti sono un elemento portatore di pace. Dove sono finiti il dialogo, l'accoglienza e la lotta al razzismo? Sono questi i valori che si insegnano oggi nelle nostre università? È inutile che ce lo nascondiamo: sono stati, sì, qualche giorno di solidarietà e di indignazione per la strage di Hamas, ma poi, improvvisamente, abbiamo assistito a un'ondata di antisemitismo, con *slogan* pro Palestina e contro Israele

altra cosa invece è offuscare gli eventi del 7 ottobre, scaricando la responsabilità su Israele, e questo purtroppo è quanto sta accadendo. Allora, visto che ci hanno insegnato che l'indifferenza

ufficialmente, in quest'Aula, una convocazione urgente, in modo che la Commissione mandi subito una lettera di stigmatizzazione nei confronti del comportamento dell'Università di Torino. Chiedo, inoltre - senza permettermi

sul Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e credo che le parole espresse dal presidente Casini su quanto sta succedendo nella Striscia di Gaza siano condivisibili;

Torino è la città antifascista per eccellenza. Torino e quell'Università sono legate da un vincolo indissolubile. A Torino si trovava il bar dove Primo Levi, Levi, Cesare Pavese e Natalia Ginzburg scrivevano le pagine più belle della Resistenza contro la dittatura. Quella non non è solo una scelta che non va bene per la ricerca italiana, che deve essere sempre protagonista: è una scelta di violenza nei confronti della storia di Torino *(Applausi)*, perché vuol dire non aver capito nulla di quello che è la città città e che rappresenta nella storia. Io, da torinese, oggi chiedo scusa a tutti quelli che hanno sempre pensato che la mia fosse una città di libertà e oggi si trovano in una città di oppressione, dove

Signor Presidente, ringrazio il presidente Romeo per avere posto nel nostro dibattito questo tema e so quanto anche il ministro Bernini sia sensibile a quanto sta avvenendo negli atenei, che - ricordiamolo hanno ovviamente autonomia e sono luoghi dove la libertà di espressione dovrebbe essere ed è particolarmente tutelata. Sono storicamente luogo di dibattito, di confronto e talvolta anche di contestazioni, che, se restano entro i binari di una dialettica politica normale, hanno caratterizzato la storia del Paese. Tuttavia, abbiamo assistito ultimamente ad effervescenze francamente difficili da sottovalutare.

a un giornalista noto per la sua competenza in temi internazionali, peraltro direttore di un giornale anche collocato, come suo diritto, in una certa galassia culturale. Nonostante questo, la contestazione è stata determinata e ha impedito l'evento. Nei giorni scorsi a Roma, all'Università

non ha avuto adeguata eco. Bisogna ringraziare il Presidente della Repubblica che ha chiamato il direttore Molinari all'indomani di quell'evento, ma c'è una situazione intollerabile di intolleranza - così va definita - molto grave. La discussione su Gaza e sul Medio Oriente dura dai tempi dell'antica Bibbia ed è più che legittima. Noi riteniamo che non si debba sottovalutare quanto sta avvenendo, tra l'altro in un combinato disposto di eventi, perché parlando sempre de «La Sapienza» c'è stata una professoressa, la De Cesare, che si è

per eccellenza della condivisione e dello scambio di idee e si trovano invece davanti il veto di prendere la parola. Ciò va condannato e penso che sia stato fatto con forza anche dalle diverse forze politiche che sono uscite apertamente. Dall'altra parte c'è però una decisione,

Capogruppo - possiamo discutere dell'ondata di antisemitismo presente in Italia. Segnalo che abbiamo anche chiesto al ministro Piantedosi, quando è venuto in audizione, di offrirci i dati,

lavorare all'interno di quella Commissione presieduta dalla senatrice Segre non per scrivere lettere o altro, ma per fare in modo che i fenomeni di antisemitismo non si diffondano. Su questo serve un'azione da parte di tutti, ma facciamo attenzione a pensare che tutto ciò che viene fatto secondo modalità che possono essere considerate a ragione di tutti democratiche sia da stigmatizzare con la stessa forza. Stiamo attenti a questo. Signora Presidente, esprimo grande perplessità e anche sconcerto, perché non capisco il motivo per cui oggi siamo qui commentare una decisione democraticamente presa all'interno del Senato accademico di un'istituzione quale quella universitaria, che giustamente di piena autonomia. Peraltro, c'è stata una votazione avvenuta a stragrande maggioranza e trovo l'ingerenza della politica particolarmente lesiva

Avanzo un'ipotesi: probabilmente ciò è anche frutto del fatto che la politica continua ad alzare i toni in maniera davvero preoccupante, alimentando scontri che, invece, dovrebbero essere tenuti a freno.

peraltro che nessuno meglio di noi possa essere considerato al corrente di come debba essere il rapporto tra il Paese, lo Stato centrale e le autonomie. Lontanissima da me l'idea di contestare la la legittimità di una decisione autonoma, ma abbiamo un sistema Paese e siamo un Paese che in questo momento si trova in una situazione complessiva in cui si deve decidere dove stare. Quello che è successo a Torino è chiaramente in contrasto con quanto la stragrande maggioranza del Paese dice e fa in questo periodo. *(Applausi)*. È chiaro

per avere sollevato la questione. Voglio sottolineare una cosa. Qualcuno ha parlato di decisione democraticamente presa: era in corso una riunione del Senato accademico, ma l'irruzione di un gruppo di studenti

Maiorino, lei è già intervenuta. Se dopo vuole intervenire per fatto personale, lo farà.

Quanto al contenuto, scrive «La Stampa» - giornale non particolarmente sospetto di essere di parte diversa da quella che è - che questo è l'antisemitismo, ossia giudicare in questo caso lo Stato d'Israele con un un metro diverso da quello che si usa per gli altri. Io non ho mai sentito parlare di interruzione dei rapporti con la Cina, che non è proprio un modello di democrazia *(Applausi)*, e ciò che succede in Tibet da decenni non è certamente una cosa lodevole, ma l'elenco potrebbe essere lungo.

emanò un regio decreto con il quale si davano agli ebrei gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini, segnando un passaggio fondamentale, perché per secoli erano stati discriminati in modo diverso nelle varie parti d'Italia che avevano diversi Governi. Il mese precedente era stata fatta la stessa cosa con i miei antenati valdesi.

studenti. Credo che abbiano il diritto di prendere la parola e dire quello che pensano: il che non vuol dire che sia giusto e bisogni giustificare tutto, ma criminalizzare l'intervento in una discussione di studenti lo trovo davvero sbagliato. Anzi, mi auguro

il decreto-legge in esame ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026; attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e della *governance* della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 SpA, statali (ANAS SpA) quale soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale, elencate nell'allegato A, e prevede che subentri alla Simico nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame. L'articolo 2 interviene sulla *governance* della Simico e, in particolare, sulle funzioni attribuite ai membri dell'organo di amministrazione. All'amministratore delegato restano attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'allegato 1, nonché per gli interventi di adeguamento delle piste da bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina e per quelli di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità «Ice Rink Oval», di Baselga di Piné. Le attribuzioni dell'organo di amministrazione in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e di rendicontazione sono delegati al consigliere di amministrazione designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che non svolge le funzioni di presidente o di amministratore delegato. Sulle funzioni delegate, l'organo di amministrazione può in qualunque momento6 impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Vengono modificate le modalità di individuazione dei due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle Regioni: mentre finora dovevano essere nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ora si prevede che uno sia designato dalla sola Regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla Regione Veneto e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Si prevede poi che sia i componenti dell'organo di amministrazione, sia quelli del collegio sindacale siano designati e non nominati e viene abrogata la disposizione che prevedeva che i componenti dell'organo di amministrazione del collegio sindacale potessero essere revocati soltanto dai soggetti che li avevano nominati. L'articolo 3 prevede che l'amministratore delegato di ANAS subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 (messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate), con i poteri di cui articolo 4, 2019, cosiddetto sblocca cantieri. L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finanziarie, mentre l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore. Gli emendamenti approvati dall'8a Commissione si concentrano, in primo luogo, sulle opere ferroviarie connesse allo svolgimento dei Giochi, prevedendo che il soggetto attuatore delle opere complementari elencate nel nuovo allegato A-*bis* sia la società Rete L'amministratore delegato di quest'ultima è nominato commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione dei passaggi a livello sulla strada statale SS 38. La società Ferrovie Nord viene invece individuata quale soggetto attuatore dell'intervento di collegamento tra il terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa e la rete ferroviaria nazionale. La Commissione ha poi previsto che l'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi tenga conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità e ha sostituito il riferimento alle Olimpiadi, presente in più punti del testo, con quello più corretto di Giochi olimpici e paralimpici. Il nuovo articolo 3-*bis*, inserito dalla Commissione, autorizza gli enti territoriali a concorrere a finalizzare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, nonché a disporre l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica, sportive e infrastrutturali, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e la funzionalità degli impianti e delle infrastrutture, nonché lo svolgimento dell'evento. Gli enti concedenti impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi sono inoltre autorizzati a procedere alla revisione del contratto di concessione, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. Si disciplina infine la destinazione delle disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'evento collaudo degli interventi, cui al piano complessivo delle opere olimpiche, e di quelle derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi. Da ultimo, si prevede che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali aggiorni gli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico. L'aggiornamento è approvato anche in più stralci funzionali, il primo dei quali riguardante il territorio Il provvedimento arriva in Aula dopo una lunga e attenta discussione in Commissione ambiente, in cui sono state svolte decine di

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Potenti.

ricordato che nel corso dei lavori in 8ª Commissione il provvedimento è stato oggetto di un approfondito esame, anche grazie all'ausilio e all'apporto di competenze professionalmente molto elevate,

nella strutturazione di iniziative edilizie in occasione di grandi eventi che, come dissi qualche giorno fa intervenendo in materia di G7, dovrebbero onorare il nostro Paese della grande

possiamo annoverare, tra gli esempi di lungimiranza, gli ammodernamenti infrastrutturali che si svolgevano nella città di Olimpia. Per diversi secoli strutture non erano adeguate ad accogliere la sempre maggior affluenza di spettatori causata dal grande e crescente interesse per quegli spettacoli sportivi. quindi una continuità nella strutturazione di opere che dovevano servire ad accogliere la massa di persone che affluivano

a momenti di totale scoramento, per noi che dobbiamo ascoltare parole di critica continua su tutto ciò che fa parte dell'esigenza di ammodernare le nostre infrastrutture. Non posso che fare riferimento, ad esempio, alle parole utilizzate nel giugno 2018 da Beppe Grillo, il quale aveva addirittura fatto un'apertura misteriosamente lungimirante alla possibilità che i suoi pargoli,

Mi domando che cosa dobbiamo fare, in alternativa, se non desideriamo ammodernare le nostre strade e le nostre ferrovie in occasione di eventi così importanti, che dovrebbero essere solo motivo di orgoglio per il nostro Paese. Invece, ogni volta diventano motivo di scontro politico e ideologico

qualche decina di chilometri di strade e realizzare due piste di atterraggio per elicotteri. Mi sembra che il parossismo arrivi a limiti inimmaginabili. Noi siamo la forza politica che spingerà il Paese e questo Governo a monetizzare le grandi disponibilità che abbiamo per realizzare le opere. Non perderemo alcuna occasione di far sì che il Paese faccia bella figura,

Governo, onorevoli colleghi, la riforma della *governance* disciplinata in questo provvedimento è dettata dalla necessità di completare le opere prima dell'evento olimpico. Del fatto che la nomina di un commissario governativo o di più commissari governativi sia la soluzione migliore mi permetto di dubitare, anche perché sono anche perché sono convinto che un commissario governativo non sia più bravo di uno nominato a livello locale. Soprattutto, nominare commissari governativi è diseducativo rispetto alla direzione che questa stessa maggioranza intende prendere con l'autonomia differenziata. Bisogna insegnare alle popolazioni ad essere autonome e non lo si fa certo mandando qualcuno da Roma che decida tutto. Permangono comunque problemi a monte, sollevati in varie sedi da diversi soggetti, anche molto qualificati, e su questi intendo soffermarmi. Cinquant'anni fa Pierpaolo Pasolini metteva in guardia sulla differenza tra sviluppo e progresso, spiegando che il primo, legato all'inarrestabile corsa a beni e profitto, non sempre portava al secondo, cioè a una crescita civile e morale, rispettosa dell'ambiente, della natura, dei territori e delle comunità che ci vivono. Quel suo scritto è di un'attualità sconvolgente rispetto a questi Giochi olimpici, raccontati e venduti come evento con ricadute positive per tutti, ma che invece ha subito dimostrato la sua insostenibilità sul piano ambientale, sociale e soprattutto economico un'insostenibilità strutturale, legata alla natura stessa di queste manifestazioni. Dalle Olimpiadi invernali del 1994 alle ultime di Pechino, tutte hanno registrato costi di gran lunga superiori a quelli preventivati: Vancouver doveva costare 2 miliardi di dollari e ne è costata 6,5; Sochi 3,5 ed ha chiuso a 9; Pechino doveva costare 4 miliardi ed è finita quasi a 10. Milano-Cortina parte da un costo di 1,5 miliardi, ma sono già stati raggiunti i 3,6 miliardi di euro. Si chiuderà a questa cifra? Chi lo sa? In ogni caso, questo grande buco verrà tappato, come al solito, con i soldi delle tasse degli italiani che le pagano. Le Olimpiadi invernali, con quella di Milano-Cortina, che non fa eccezione, hanno peraltro smesso da decenni di produrre valore a livello locale, ma riflettono, a pieno titolo, un approccio predatorio ai territori, che vengono piegati alle logiche del *business*, del cemento e dell'asfalto, nonché a quello della diffusione delle immagini dell'evento, con poca o nulla attenzione rispetto alle ricadute ambientali o alle reali necessità delle popolazioni di montagna. popolazioni avrebbero bisogno oggi di essere sostenute in quanto garantiscono i servizi ecosistemici, la protezione della biodiversità e il mantenimento degli equilibri ambientali. Forse che i soldi dei giochi verranno destinati almeno in parte a servizi sanitari, a quelli educativi o a forme di trasporto pubblico più efficienti per gli abitanti della montagna? Direi proprio di no.

strizzando l'occhio alle imprese che ne trarranno lavoro e guadagno. A parte il fatto che le infrastrutture andrebbero fatte tutte le volte che ce n'è bisogno e non solo in occasione di un grande evento, la sola vicenda della pista da bob dimostra come questa argomentazione sia falsa e fuorviante.

81 milioni e rotti di soldi pubblici spesi per un impianto che avrebbe forse senso fare a 2.500 metri, ma non certo a 1.300, senza neppure la certezza di farcela in tempo. Un'opera bandiera, ma insostenibile, visto che in Italia appena 59 persone praticano questo sport. Considerato inoltre che le temperature saranno sempre più alte mantenere l'impianto costerà sempre di più, ben oltre la cifra stimata di diverse centinaia di migliaia di euro all'anno, che è comunque enorme e a carico del Comune, quindi della popolazione locale. ampia però è la questione della sostenibilità ambientale ed economica. Il cambiamento climatico ha fatto ammalare la montagna, che è sempre più fragile e sempre meno in grado di reggere la costruzione di opere invasive. Guarda caso, invece, per queste Olimpiadi vengono realizzate opere che per la gran parte sono arterie stradali, spesso sovradimensionate rispetto alle necessità effettive dei territori, che richiederanno nel tempo grandi spese di manutenzione. strade, gallerie e ponti hanno alti costi di manutenzione. In Italia abbiamo tristi esperienze recenti dei disastri che possono accadere quando le manutenzioni non vengono fatte, oltre al fatto poi che si tratta di opere finalizzate a una mobilità inquinante e vecchia, quella del trasporto pubblico su gomma. La mobilità *soft* rientra però nell'ideologia *green* che va combattuta, perché così vogliono le *lobby* amiche del nostro Governo una figuraccia internazionale annunciata per l'Italia, che sottolineerà ulteriormente la nostra triste nomea di Paese cicala, sprecone e canterino. Nondimeno, queste Olimpiadi rischiano di danneggiare anche la città di Milano, facendo ulteriormente esplodere i prezzi delle case nelle zone adiacenti al villaggio olimpico, con l'effetto di espellere gradualmente gli attuali residenti e restringendo ulteriormente il diritto all'abitare delle fasce più deboli. Non avrebbe avuto più senso riqualificare le strutture esistenti, come il vecchio Palasport di Milano? Perché questo spreco in una fase di contrazione della spesa pubblica per opere che andranno solo ad acuire vecchi e nuovi problemi? Soprattutto, che fine ha fatto l'impegno per Olimpiadi sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, peraltro firmato? Quando le proteste sono così trasversali, quando sono in grado di unire la montagna e una città come Milano, significa che la questione è molto seria e non può essere liquidata con un'alzata di spalle, parlando dei soliti professionisti del no. Le iniziative di protesta stanno invece ponendo una questione essenziale, essenziale, che riguarda il nostro futuro e i nostri modelli di sviluppo che queste Olimpiadi non vedono, chiuse come sono in una lettura antiquata e superata del mondo, quella che, per tornare a Pasolini, insegue lo sviluppo senza rendersi minimamente conto che questo non porterà alcun progresso, ma semmai il contrario.

quando ci si appresta a fare grandi eventi, bisogna sempre mettere sul piatto della bilancia gli elementi positivi, come il fatto che il nostro Paese sarà trasmesso sulle televisioni di tutto il mondo per molti giorni, e gli aspetti negativi, come riuscire a contemperare le grandi infrastrutture che si stanno realizzando con l'ambiente e la società circostante.

a un certo punto ha deciso di non partecipare a quelle Olimpiadi, una scelta nefasta perché noi le infrastrutture, a differenza di Milano e di Cortina, ce le avevamo già, ed erano quelle delle Olimpiadi del 2006.

ma è stata fatta una scelta demagogica da parte dell'amministrazione e quelli che sono venuti dopo, il sindaco Lo Russo e il presidente Cirio, nulla hanno potuto fare per recuperare una situazione compromessa, in parte anche grazie alla non grande collaborazione delle due città, che, una volta appropriatesi delle Olimpiadi e dei finanziamenti, non sono state così generose da far rientrare chi si era autoescluso.

l'ambientalismo e la decrescita e non si percepisce la possibilità di cambiare la storia. La mia città nel 2006 ha radicalmente cambiato faccia:

nel quartiere Lingotto e quindi quella fabbrica ce l'avevo ben presente. E invece Torino è diventata una città turistica e oggi le persone che vi arrivano non trovano più la città fabbrica, ma trovano una città

esattamente come prevedevamo noi nel nostro piano *shock*, ci vogliono commissari *ad hoc*. Spero che le comunità vengano ascoltate

perché sicuramente il Veneto produttivo non ha infrastrutture così adeguate. La Milano produttiva sta meglio di altri, ma non è così servita al di fuori della cerchia cittadina, quindi probabilmente questo

per una pista o per qualsiasi altro elemento. Questo è un rammarico doppio: per la mia città, perché avrebbe fatto bene al suo PIL e al suo indotto, e per la collettività italiana, che vede sprecate risorse che evidentemente si potevano utilizzare per far altro, di cui questo Paese ha drammaticamente bisogno. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il primo *question time* di questa legislatura si è svolto quasi un anno e mezzo fa con il ministro per lo sport e i proprio sulle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ricordo bene quel momento, perché è stato anche il mio primo *question time* e in precisazioni riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica di quei giochi invernali. Un anno e mezzo fa, il ministro Abodi ci assicurò che si sarebbero seguiti tutti i principi e i criteri ambientali richiesti dal Comitato olimpico internazionale e garantì che avrebbero rispecchiato i valori e la volontà esplicita della Fondazione

si è intestardito nel voler portare il progetto della pista da bob a Cortina, questa volta definita in versione *light* - o pseudo-*light*, perché comunque costerà lo stesso 122 milioni di euro - sacrificando centinaia di larici secolari. Si è anche deciso di fare di più, cioè di asfaltare e costruire strade a più non posso in mezza Italia del Nord, già intasata dal traffico e dall'inquinamento atmosferico. Tutto questo per la modica cifra di 3 miliardi di euro, per far fare bella figura all'Italia, come pensa il ministro Salvini, mentre stiamo facendo una figuraccia planetaria, con buona pace della sostenibilità, ma con il benestare del presidente leghista del Veneto Zaia, che, sempre a parole, aveva inizialmente dichiarato che queste Olimpiadi sarebbero state ad impatto impatto zero. Purtroppo non sarà così, ma poco importano le parole di ieri, tant'è che oggi arriviamo a discutere il decreto-legge recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della società Simico, in un contesto in cui nel frattempo gli effetti della crisi climatica avanzano e con essi anche le criticità legate alla carenza di neve, che stanno preoccupando il settore del turismo invernale, la sua economia e anche il circo bianco. Ciò che importa alla Regione Veneto e al Governo è la pista da bob di Cortina, una vicenda che ha assunto contorni assurdi e inaccettabili, anche per la palese incompetenza con cui quest'opera viene gestita, rischiando che rimanga una carcassa inutilizzata, visti i tempi ristrettissimi per la sua realizzazione. è di più. Nell'ulteriore tappa del percorso ad ostacoli di queste Olimpiadi, il Governo sta continuando ad accumulare enormi ritardi nella realizzazione di opere e infrastrutture, tra sprechi e incalcolabili danni ambientali. È una faccenda che ha del grottesco, ma fa anche arrabbiare, olimpico internazionale (COI) nell'organizzazione dell'evento olimpico ha chiesto il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e ha optato per il nostro Paese proprio per l'attenzione manifestata dai proponenti italiani nel *dossier* di candidatura alla tutela paesaggistica e ambientale dei luoghi coinvolti nello svolgimento delle gare: una vera beffa e anche una presa in giro,

pertanto, a meno di due anni dall'inizio dei giochi, ci troviamo a modificare, con questo decreto-legge, le funzioni attribuite all'organo di amministrazione di Simico, per cercare di supplire alla difficoltà gestionale di questa società. Inoltre, in merito all'improvviso cambio di *governance* all'interno di Simico, ci stupisce che sia stato possibile affidare la sua gestione all'ingegnere Sant'Andrea, sostituito giusto poche settimane fa da un nuovo commissario, dopo che lo stesso Sant'Andrea, anche in occasione della Campionati del mondo di sci a Cortina, aveva lasciato il proprio incarico di commissario alcuni mesi prima delle gare, anche in quel caso ad opere incompiute. Oggi, come allora, stesso copione. A fronte di queste notizie, che francamente ci preoccupano, il decreto-legge oggi in discussione tenta di mettere una toppa alla mala gestione di Simico, affidando la realizzazione delle opere stradali connesse allo svolgimento delle Olimpiadi ad ANAS. ad ANAS. Per noi di Alleanza Verdi e Sinistra però questa delega ad ANAS è molto preoccupante, perché ci si concentrerà esclusivamente sulla realizzazione di opere stradali verranno bypassati la valutazione del rischio idrogeologico, il principio di sostenibilità ambientale e gli sforzi che vanno fatti per potenziare una mobilità sostenibile oggi più che mai necessaria. Il passaggio ad ANAS evidenzia anche le forti criticità in materia di tempistiche. La promessa che le opere saranno terminate per l'inizio dei giochi invernali si sta rivelando un miraggio. Si rischia di non vedere il completamento delle opere già in cantiere,

ormai da troppo tempo dalla Lega. Questo grande evento doveva consentire il potenziamento di importanti tratte ferroviarie tra la Lombardia e il Veneto, che per più della metà sono sotto il livello minimo di soddisfacimento. Non vi nego la mia incredulità nel venire a sapere dal sindaco di Bergamo Gori che non si riusciranno a completare nemmeno i 6 chilometri di ferrovia necessari per collegare l'importante scalo aeroportuale di Bergamo Orio al Serio alla stazione dei treni già predisposta per le Olimpiadi, ma che non sarà pronta per l'inizio delle gare. Stesso destino per l'aeroporto di Verona, che avrebbe dovuto collegare la stazione ferroviaria della città. Non si è nemmeno collegato e completato l'anello ferroviario delle Dolomiti, un progetto fortemente sostenuto dai cittadini, ma che sembra naufragato nel nulla. Nel complesso, per la rete stradale italiana si spenderanno 3 miliardi di euro e solo 400 milioni per la mobilità ferroviaria, sempre che si riesca a completarla. In audizione ci hanno detto che non c'è più tempo per iniziare o ultimare le tratte ferroviarie: questa è la litania che abbiamo sentito in audizione. Solo che sono passati anni dall'annuncio dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina e ha dell'incredibile che tali opere non siano state programmate per tempo e che non siano neanche state iniziate. Nel nostro lavoro emendativo abbiamo chiesto di valutare l'impatto ambientale per le opere di Milano-Cortina 2026, mentre per la mobilità su rotaia abbiamo presentato un emendamento che prevede la nomina di un commissario straordinario per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie, finanziati per i Giochi. Amareggia molto sapere che le conseguenze di questa politica retrograda graveranno sul presente e sul futuro dei nostri ragazzi, sulle intere comunità che ci vivono e sui luoghi di inestimabile valore ambientale e paesaggistico che abbiamo la fortuna di avere. In tutto il lavoro che sto svolgendo da un anno e mezzo a questa parte per Milano-Cortina un lato positivo c'è, che dà anche un minimo di sollievo, ed è sapere che le comunità montane, i territori montani associazioni, come Mountain Wilderness, Italia Nostra e altre, lasciati soli ad affrontare le difficoltà quotidiane, non si arrendono di fronte al *modus operandi* inaccettabile e arrogante della classe politica dirigente. A loro vanno il mio sostegno, la mia voce e il mio ringraziamento per l'immane lavoro che stanno svolgendo a tutela del nostro territorio, perché è anche nostro. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra non diciamo «no»

che spreca soldi pubblici, deturpa l'ambiente e non garantisce nemmeno uno svolgimento sicuro dei giochi, né di terminare in tempo le opere previste, ma fa fare all'Italia una figuraccia a livello internazionale.

non è la prima volta in quest'Aula, è la prima volta da questo scranno, che fu del mio grande amico e maestro, la persona che mi ha cambiato la vita, il presidente Silvio Berlusconi. Al suo fianco, ho condiviso per oltre quarant'anni, come noto e come lei sa, Presidente, la vita, il lavoro e la grande passione non solo per il calcio, ma per tutto ciò che è sport. Ricordo che il presidente Berlusconi mi diceva che lo sport in generale e il calcio afferiscono alla sfera non del *business*, ma dei sentimenti, e assomigliano un po' alla religione, con i suoi misteri dolorosi e gaudiosi. Così siamo sempre andati avanti insieme, passando da Istanbul ad Atene, dall'eliminazione con il Cittadella alla vittoria con il Pisa, la con conseguente promozione in serie A per la prima volta del Monza. Da uomo di sport, sono molto felice e orgoglioso che l'Italia ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. Come diceva il presidente Berlusconi, lo spirito olimpico di De Coubertin conferma il valore dello sport ed invita a superarsi lealmente. La mia passione per lo sport ho cercato di dimostrarla da subito, anche in questo consesso, sostenendo attivamente il percorso che, partendo dalla passata legislatura, ha portato all'inserimento dello sport in Costituzione. In tal senso, ho già presentato in questa legislatura un nuovo disegno di legge che punta proprio all'attuazione di quell'articolo 33 della Costituzione che mira a migliorare il sistema sportivo in Italia, soprattutto in ambito formativo e di accesso alle pratiche e agli impianti per i soggetti che hanno maggiori difficoltà ad integrarsi. È sicuro che lo sport è un elemento fondamentale per ogni società. Intervengo dunque su un argomento che mi è particolarmente caro, le Olimpiadi, che si svolgeranno anche nel territorio in cui sono nato, cresciuto ed eletto, vivo e ho sempre svolto le mie attività: la Lombardia. Ricordiamo tutti le tristi immagini delle strade delle nostre città vuote, con le attività completamente ferme e uno stravolgimento totale delle nostre vite. In termini assoluti, la città in cui il conto del Covid è stato più alto è appunto Milano, con oltre 650 milioni di euro Oggi dunque le Olimpiadi invernali Milano-Cortina rappresentano una linfa nuova di sviluppo. I lombardi, gente laboriosa e produttiva, hanno già affrontato in maniera eccelsa la ripresa dalle varie crisi che si sono succedute nel tempo ed oggi sono pronti a mettersi in gioco per dare al mondo un evento grandioso, con la convinzione di superare tutte le aspettative. Le Olimpiadi sono un evento che coinvolge tutto il comparto sportivo e non solo, dagli atleti in campo agli allenatori, agli organizzatori, ai volontari, alle istituzioni del territorio ed agli imprenditori. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono la quarta Olimpiade che il nostro Paese ospita, un dato molto importante. Le medaglie olimpiche, in ricordo delle precedenti edizioni che l'Italia ha ospitato, sono conservate nella sala del Consiglio dei Ministri, a dimostrazione dell'importanza che le Olimpiadi hanno per la nostra identità e per la nostra storia. Inoltre, questa manifestazione sarà senza dubbio un volano per l'intera economia nazionale. Ci sarà un aumento della domanda per il comparto sport che potrebbe superare il miliardo di euro

Secondo la ricerca di una prestigiosa università romana, la sola organizzazione delle Olimpiadi invernali può produrre nel sistema Paese quasi 13.000 nuove unità di lavoro, oltre 9.000 delle quali per il settore sportivo e quasi 4.000 per i settori economici ad esso collegati. I benefici non si limiteranno però agli aspetti economici: non sottovalutiamo l'impatto mediatico di un evento di questa portata, che potrebbe invogliare sempre più persone ad avvicinarsi alla pratica sportiva nel nostro Paese. Pur attestandoci sotto la media europea, i cittadini italiani che praticano sport in modo continuativo sono in media aumentati, dal 22,8 per cento del 2010 al 27,1 del 2020, un dato che potrebbe continuare Si pensi, ad esempio, all'impatto dei successi nel tennis di Jannik Sinner e della Nazionale che ha conquistato l'ultima Coppa Davis. Secondo la Federazione italiana tennis e padel, infatti, il numero di tesserati è passato da 129.000 nel 2021 a 660.000 nel 2023, ma le stime indicano oltre 700.000 tesserati all'inizio del 2024. Anche il numero di praticanti è aumentato in modo considerevole, passando da circa 1,3 milioni nel 2021 a 4,5 milioni nel 2023, per non parlare degli effetti economici estremamente positivi derivanti dall'aumento degli spettatori, dei turisti e degli investitori stranieri collegati al mondo del tennis. Lo sport riveste un ruolo sociale di grande rilevanza, che garantisce significativi effetti positivi, non solo materiali, per la nostra società. Si pensi al miglioramento del benessere psicofisico, all'incentivo alla coesione sociale, alla riduzione della spesa sanitaria e alla promozione del territorio. Dunque queste Olimpiadi per l'Italia hanno un'enorme importanza, *in primis* per l'orgoglio che saranno capaci di imprimere nel nostro Paese e per l'effetto dirompente che avranno per l'intera economia, per il comparto sport e per la società italiana tutta. È innegabile dunque che l'effetto di questo provvedimento, che oggi ci accingiamo a votare, sarà la sicura modernizzazione dei territori coinvolti. Le nuove infrastrutture faciliteranno le comunicazioni e renderanno il Nord Italia ancora più competitivo, il tutto garantito da una *governance* efficace e snella, che il Governo si è impegnato ad attuare. È importante quindi il coinvolgimento di tutti gli enti, delle organizzazioni e delle associazioni del territorio, che saranno in grado di dare la giusta collaborazione per il perfezionamento di questo evento. Facciamo sì che le infrastrutture che nasceranno non siano finalizzate alla sola manifestazione, ma diventino luoghi di aggregazione e partecipazione anche per il futuro. Cari colleghi, il nostro partito, com'è noto a tutti, è sempre favorevole all'organizzazione di grandi eventi pubblici, in particolare di grandi eventi sportivi come le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali. Credo quindi che questa manifestazione debba essere assolutamente sostenuta e amministrata nel miglior modo. Il Governo è impegnato in prima linea per rendere un successo le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e noi saremo al suo fianco.

rappresentanti del Governo, questo provvedimento, al pari di altri proposti da questa maggioranza, non è altro che fumo negli occhi, perché non risolve e non affronta i temi e i problemi che restano sul tavolo. Per restare in tema - mi con questo provvedimento sparate a pieni cannoni neve artificiale sulla vostra incapacità di investire e spendere soldi provenienti dalle casse dello Stato, quindi dalle tasche dei cittadini. Nel corso delle audizioni in Commissione, sia le associazioni di categoria sia i rappresentanti degli enti locali hanno sollevato non poche perplessità sulle previsioni di questo decreto-legge, ma con voi - si sa - è inutile cercare un confronto. La quasi totalità degli emendamenti correttivi e integrativi che il mio Gruppo parlamentare ha proposto aveva lo scopo di migliorare il testo, ma ovviamente sono stati respinti, dietro un parere contrario del Governo. Si trattava di interventi di buon senso, mirati appunto a rendere efficace e propositivo un testo completamente lacunoso. Prima di ogni cosa, mi preme sottolineare, com'è già stato fatto dalla collega Floridia, che questo testo non tiene davvero conto, in alcun modo, della vocazione sostenibile

Pensiamo alla famigerata pista da bob: già nel mese di dicembre un cospicuo gruppo di colleghi, tra cui anche diversi parlamentari del MoVimento 5 Stelle, si rivolsero al Comitato olimpico internazionale e alla Presidente della Commissione di coordinamento per i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, chiedendo di intervenire nella scelta del luogo già individuato per l'edificazione della In quell'occasione, in sostanza, si chiedeva di indicare una sede già esistente, ma fuori dall'Italia, secondo i criteri di sostenibilità assunti dall'Agenda olimpica 2020 per lo svolgimento delle gare da bob, viste la ristrettezza dei tempi per la realizzazione della pista e l'assenza di alternative; e invece no, per voi è tutto regolare (come si suol dire, va tutto bene, madama la marchesa). Non vi siete fermati neanche di fronte all'abbattimento di centinaia di larici secolari che dovranno far posto a questa pista da bob, impattante

e anche dei cittadini e del territorio, si è dovuto arrendere, constatando che la tutela dell'ambiente di certo non è musica gradita a questo Governo. Noi del MoVimento 5 Stelle, come dicevo poco fa, abbiamo provato a cambiare questo testo e a migliorarlo. Ad esempio, abbiamo proposto l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la manutenzione e la sicurezza di strade, ponti e viadotti. Abbiamo anche chiesto - ma non ottenuto, ovviamente - l'ammodernamento del trasporto pubblico locale attraverso l'acquisto di una nuova flotta di autobus con emissioni rientranti nei limiti Euro 6. ci avete accontentato con l'accoglimento di ordini del giorno, ma sempre con la solita formula edulcorata: a valutarne l'opportunità, entro i limiti della finanza pubblica. Poca roba, insomma. Sono impegni che, sì, assumete, ma che, nella chiara prospettiva della manutenzione di strade e opere d'arte già esistenti e del rinnovo di flotte di autobus obsolete e inquinanti in un'area che è la più inquinata d'Italia, sono e resteranno impegni al ribasso, di cui lascerete traccia solo sulla carta. Ancora, per assicurare la massima trasparenza e il monitoraggio delle opere abbiamo proposto di trasmettere anche al Parlamento

di denaro pubblico da voi previsto per rimborsare il commissario e i suoi subcommissari. Abbiamo provato a ridurlo a 20.000 e anche chiesto di azzerarlo. È un commissario straordinario che forse voi vorreste in eterno, i cui poteri invece dovrebbero, a nostro avviso, esaurirsi con l'avvio dei Giochi, ma anche questi semplici concetti sono quanto di più lontano dalle vostre politiche. Nel nostro Paese, l'emergenza rappresentata dalla sicurezza sui luoghi di lavoro viene presa in considerazione

ma, anche in quest'ultimo caso, per voi va tutto a gonfie vele. Avete bocciato la nostra proposta per tutelare gli operai impiegati nei luoghi

Quando si prevede di realizzare grandi opere in un lasso di tempo molto breve, ciò che viene da immaginare è lo *stress* al quale possano essere sottoposti gli operatori dei cantieri, con lavori da svolgere senza soluzione di continuità, come riferito in audizione, in orari notturni e diurni. Per voi però va bene così, sordi come siete alle richieste di maggiori tutele per i lavoratori e di maggiore sicurezza avanzate, da ultimo e in maniera più frequente, anche dal presidente Mattarella. Bocciato anche il finanziamento del fondo per le reti ciclabili urbane: la cosa non ci stupisce affatto, perché un ciclista è è un disastro per l'economia del Paese; non compra auto, quindi non prende soldi in prestito per acquistarne, non paga polizze assicurative, non compra carburante, non paga per sottoporre l'auto alle necessarie manutenzioni e riparazioni, non utilizza parcheggi a pagamento, non causa incidenti rilevanti, non richiede autostrade a più corsie e non diventa obeso. Le persone sane non sono necessarie, né utili all'economia: non comprano medicine e non vanno negli ospedali, né dai medici. Non aggiungono nulla al PIL del Paese. Questo non lo dico io, ma lo ha detto un banchiere, uno dei vostri cari amici, davanti a una platea di economisti, ed evidentemente li ha fatti molto riflettere. A tal proposito, colleghi, parlando di amici, avete visto gli ultimi dati sugli utili delle banche? Quasi 24 miliardi. Ma guardiamoci intorno: in Spagna hanno avuto il coraggio che a voi è mancato e la tassa sugli extraprofitti delle banche ha portato nelle casse dello Stato un miliardo di euro. Pazienza, è tutto nella norma. Signor Presidente, concludo ribadendo che questo provvedimento manca di concretezza ed incisività. In estrema sintesi, è lo specchio del vostro modo di guidare il Paese.

l'Italia arriva ad ospitare, nel 2026, uno degli eventi sportivi più importanti. Le Olimpiadi sono un momento straordinario di partecipazione e di coinvolgimento. Arriveranno a far partecipare tutti i Paesi del mondo, aprendo così una grandissima vetrina e anche un *monitor* su tutta l'Italia, dando la possibilità non solo di vedere una competizione sportiva che appassiona tutti e unisce tutti i popoli, ma anche la possibilità di vedere l'Italia

al limite e di veramente diabolico. Questa sfida, la sfida delle Olimpiadi, ci vede pronti però e l'Italia è pronta.

Queste Olimpiadi noi le vediamo solo ed esclusivamente perché ci sono state due Regioni e due presidenti di Regione, che si chiamano Luca Zaia e Attilio Fontana, che le hanno fortemente volute. grazie alla partecipazione delle Regioni si è riusciti ad arrivare all'approvazione della nostra candidatura; questo non sarebbe accaduto, se non avessimo avuto il ministro Giancarlo Giorgetti *(Applausi)*, che al tempo, con la delega allo sport, ha fortemente combattuto, ponendosi a fianco delle Regioni

lo sviluppo infrastrutturale e il rafforzamento dell'immagine dell'Italia all'estero. Il decreto-legge in esame prevede una serie di misure volte a revisionare le attribuzioni commissariali e a riformare la *governance* della società. un decreto, però, che - dobbiamo dirlo con onestà - certifica e rende palese il fallimento del Governo di molte Regioni, anche di quelle ricordate prima dalla collega, prima dalla collega, nel far fronte agli impegni assunti, come il fallimento dei mirabolanti annunci del nuovo codice degli appalti, che avrebbe dovuto risolvere qualsiasi problema, mentre tutte le volte non si trova in grado di far fronte alle necessità del Paese. È a causa di questi fallimenti che il decreto-legge oggi in esame deve adottare misure straordinarie per accelerare i lavori, per garantire che tutte le infrastrutture necessarie siano pronte in tempo utile per i Giochi. Certificate e chiarite le responsabilità del Governo, però, come senatori del Partito Democratico, riteniamo comunque nostro dovere assicurare il successo dell'evento, così come riteniamo al contempo imprescindibile che tutte le opere infrastrutturali e accessorie siano realizzate nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e sostenibilità, per lasciare un'eredità duratura al nostro Paese e alle generazioni future. La discussione di oggi rappresenta dunque un momento di riflessione per valutare attentamente le disposizioni previste, esprimere le nostre considerazioni e contribuire, ognuno secondo le proprie convinzioni, al perfezionamento di un provvedimento di tale rilevanza. Lo premetto e lo ribadirò: condividiamo l'obiettivo di garantire all'Italia di essere pronta ad accogliere uno degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti a livello internazionale. I Giochi olimpici e paralimpici invernali rappresentano infatti un'opportunità unica per il nostro Paese di mostrare al mondo le nostre capacità organizzative, la nostra cultura sportiva, cultura sportiva, le bellezze naturali e architettoniche che rendono l'Italia unica. Tuttavia, pur riconoscendo i giusti obiettivi perseguiti, non possiamo trascurare di evidenziare alcune preoccupazioni che ci spingono a una posizione di cautela. Dalla nostra analisi del testo e dalle audizioni realizzate emergono infatti preoccupazioni riguardanti principalmente la trasparenza nelle procedure di affidamento, la qualità delle opere, l'impatto ambientale dei progetti infrastrutturali e la reale distribuzione dei benefici economici tra le comunità locali. In primo luogo, il trasferimento di competenze all'ANAS, pur essendo una mossa volta a snellire i processi burocratici, solleva questioni importanti riguardo alla trasparenza e alla concorrenza nell'assegnazione dei lavori, mentre l'accelerazione dei lavori, se è indubbiamente necessaria per rispettare i tempi previsti, non deve avvenire a discapito della qualità degli interventi. Infine, è fondamentale che i benefici economici generati dall'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici siano distribuiti equamente, portando a un vero sviluppo delle comunità locali. Le modifiche alla *governance* della società e l'accentramento di alcune funzioni potrebbero invece rischiare di escludere dal processo decisionale le realtà locali che dovrebbero essere coinvolte attivamente per per assicurare che le opere realizzate rispondano alle esigenze del territorio e contribuiscano allo sviluppo sostenibile delle Regioni ospitanti. Queste preoccupazioni, onorevoli colleghi, ci portano a richiedere un approfondimento su vari temi. È nostro dovere garantire che un evento di tale importanza sia un'opportunità di crescita non solo economica, ma anche sociale e ambientale.

proposte di modifica sono state oggetto di emendamenti del nostro Gruppo, parte dei quali è stata approvata grazie al proficuo lavoro svolto come sempre in 8a Commissione e al dialogo avvenuto in questa occasione con il Governo Fra questi emendamenti sottolineo un'attenzione non solo ai collegamenti stradali, ma anche a quelli ferroviari, con l'individuazione di Ferrovienord quale soggetto attuatore dell'importante intervento per il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Malpensa e, a seguire, l'emendamento per consentire agli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici di concorrere a finanziare e a svolgere attività inerenti

Avremmo auspicato la sua approvazione in Commissione, ma vogliamo dar credito all'impegno del Governo di perseguirne comunque le finalità; impegno che si è preso accogliendo l'ordine del giorno in cui sono confluiti i contenuti del nostro emendamento. Dobbiamo al contempo evidenziare che sono state invece respinte le tre proposte contrarie alla revisione della *governance* e al funzionamento della Società Infrastrutture Milano-Cortina 2016, di cui non si comprende la finalità, se non quella di sostituire il vertice manageriale, e le proposte volte a limitare i rimborsi per lo svolgimento delle funzioni commissariali poste a carico delle risorse per realizzare le opere. Alla luce di questo dialogo e di questa collaborazione su alcuni aspetti, ma anche delle chiusure su altri altrettanto rilevanti, possiamo quindi concludere la nostra valutazione ribadendo la nostra attenzione all'importanza strategica dei Giochi olimpici e paralimpici invernali per l'Italia, non solo in termini di visibilità internazionale, ma anche per le opportunità di sviluppo economico, sociale e infrastrutturale. Tuttavia, le preoccupazioni sollevate in merito alla trasparenza delle procedure di affidamento, alla sostenibilità ambientale dei progetti, al coinvolgimento delle comunità locali e all'equa distribuzione dei benefici economici, ci spingono a chiedere ulteriori riflessioni e miglioramenti al testo. Abbiamo proposto modifiche concrete con l'intento di rendere il decreto-legge più inclusivo, trasparente e attento

È opportuno ricordare le premesse su cui poggia il provvedimento in esame e che ritroviamo nel decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale venivano introdotte disposizioni urgenti - lo sottolineo - già nel 2020 per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e si identificava la Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni Lombardia e Veneto, nonché dalle Province autonome di Trento e Bolzano, quale soggetto che doveva occuparsi della progettazione, nonché della realizzazione, in quanto centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche.

26 settembre 2022 l'allora presidente del Consiglio Draghi approvava il piano degli interventi. Il complesso di interventi quota circa 3 miliardi di euro per circa 110 interventi infrastrutturali. Era necessario dare queste informazioni, seppur sommarie, perché in questo modo emerge con chiarezza che le opere da realizzare, tranne qualche modifica davvero lieve, sono state individuate ed approvate dagli scorsi Governi. In altre parole, la programmazione degli eventi è stata decisa anche con l'appoggio di chi oggi critica il provvedimento in discussione provvedimento che, nei fatti, non fa altro che imprimere un'accelerazione alla realizzazione delle opere, prevedendo il passaggio dalla Società infrastrutture Milano-Cortina 2026 ad ANAS del ruolo di soggetto attuatore di alcune opere di impiantistica sportiva e infrastrutturale, stradale e ferroviaria e il subentro nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla medesima società, il tutto nell'ambito degli accordi quadro con ANAS, che consentono di procedere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure ad evidenza pubblica.

Questa scelta è stata salutata positivamente da tutte le istituzioni coinvolte, poiché consente un'accelerazione effettiva alla realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento delle Olimpiadi. Mi permetto di richiamare un esempio per tutti, ossia il caso portato dal sindaco di Lecco, sentito in audizione in 8a Commissione, il quale ha sottolineato che grazie al passaggio di competenze ad ANAS verrà inaugurato a breve il tratto di strada Milano-Bormio verso Lecco, che consiste in un ponte che attraversa l'Adda. Anche la revisione della *governance* della società, contenuta nel provvedimento oggi in discussione, è finalizzata alla necessità di assicurare una gestione più efficace che si raccordi meglio con il passaggio di competenze ad ANAS,

Nonostante si tratti di norme di buon senso, l'opposizione - come abbiamo sentito tutti - critica strumentalmente questo decreto-legge, come all'epoca lo stesso MoVimento 5 Stelle criticava la scelta di appoggiare la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi. Al di là del prestigio per il nostro Paese di ospitare le Olimpiadi invernali, la lettura di qualche dato riguardante l'importanza strategica di questo evento può aiutarci a fare riflessioni più accurate. Le ricadute economiche delle Olimpiadi del 2026 sui territori sono valutate, da tre differenti studi condotti dalle università La Sapienza di Roma, Bocconi di Milano e Ca' Foscari di Venezia, in circa 4,5 miliardi di euro, euro, al netto degli investimenti per la realizzazione del grande evento. Secondo lo studio realizzato dall'università Ca' Foscari di Venezia, i posti di lavoro generati dall'evento sarebbero 13.800 per le sole Regioni Veneto e Trentino, senza contare la Lombardia. Eppure, come dicevo, c'è chi fa ostruzionismo. È ovviamente un ostruzionismo di facciata, ideologico e senza senso; il tipico ostruzionismo che si fa perché va fatto e perché non farlo significherebbe ammettere che questo Governo sta facendo bene. Ciò è accaduto ad esempio anche per le opere relative agli eventi legati al G7. Stiamo parlando dell'opposizione a un provvedimento che è priva di fondamento, un no che non sarà il primo e non sarà neanche l'ultimo. Vorrei ricordare a quest'Assemblea che il 10 gennaio 2019, quando il Consiglio dei ministri ha garantito il sostegno alla candidatura di Milano e Cortina, il presidente era Giuseppe Conte. Il 24 giugno 2019 a Losanna il COI ha designato vincente la candidatura candidatura Milano-Cortina e, durante la presentazione finale, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha confermato il pieno sostegno al progetto olimpico. Oggi però assistiamo all'ennesimo teatrino del no: le opere non vanno bene; l'impatto ambientale non è stato valutato; costa troppo. Coloro che oggi criticano questo provvedimento, che non modifica assolutamente il progetto originario, ma cerca di accelerare la realizzazione delle opere, ieri hanno votato i provvedimenti che ne gettavano le basi. Non è davvero possibile credere che solo oggi vi ricordiate dell'impatto ambientale, facendo finta di non sapere che, prima della realizzazione, ogni opera dev'essere sottoposta a tutte le valutazioni e autorizzazioni ambientali previste dalla legge. La stessa cosa vale per le norme sulla sicurezza del lavoro, cui nessuno può sottrarsi. Solo per essere chiari nei confronti dei cittadini, la tanta criticata pista di bob di Cortina, che per l'opposizione è inutile e dannosa per l'ambiente, sarà la prima infrastruttura sportiva al mondo ad ottenere la certificazione Envision, la certificazione di qualità delle infrastrutture più completa che ad oggi sia possibile ottenere. Basti pensare che la certificazione Envision analizza l'opera sotto il profilo dell'efficacia dell'investimento, del rispetto dell'ecosistema, del rischio climatico e ambientale, della durabilità della *leadership* e del miglioramento della qualità della vita. In particolare, il protocollo innovativo valuta le *best practice* che un progetto infrastrutturale dovrebbe mettere in atto nell'approcciarsi all'ambiente e al mondo naturale, sotto il profilo dell'impatto sia paesaggistico sia sulla biodiversità e sugli equilibri idrici esistenti. La famigerata pista da bob, che sarà in parte bonificata e in parte recuperata e migliorata, costituirà un fiore all'occhiello per Cortina. Ancora, si insiste sul fatto che sarà il Comune a dover sostenere le spese di gestione della pista. Evidentemente, le audizioni in Commissione non servono a nulla, perché, su esplicita domanda, la Vice Presidente della Regione Veneto ha già chiarito che la gestione sarà a carico della Provincia di Trento e Bolzano, delle federazioni sportive e della Regione Veneto. È evidente a questo punto perché i partiti del "no a prescindere" non possano trovare spazio in Italia, che ambisce a incrementare le sue potenzialità e a creare sviluppo e lavoro. È altrettanto evidente perché risultino infondate tutte le eccezioni contro questo provvedimento, provvedimento, che, come ho più volte ribadito, sono dettate dal solo fatto di essere opposizione e nel solo tentativo di esercitare un qualche ruolo. In definitiva, con questo provvedimento il Governo Meloni punta a chiudere il *dossier* Olimpiadi in tempo, affinché tutto il mondo possa ammirare quanto l'Italia ha da offrire in termini di sport invernali e non solo.

come sapete, oggi ricorre il trentesimo anniversario dell'assassinio della giornalista del TG3 Ilaria Alpi Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin, avvenuto a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Ilaria e Miran si trovavano in Somalia per seguire giornalisticamente una pista su degli ignobili traffici clandestini di armi e tangenti e proprio quella pista, purtroppo, fu per fu per loro fatale. Quel giorno un commando aprì il fuoco su di loro prima di fuggire via. Da allora è iniziata una lunghissima vicenda processuale senza che mai si riuscisse a fare del tutto piena luce su questa vicenda. Gli assassini materiali e i loro mandanti, ancora oggi, sono ignoti:

Come ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, le medaglie d'oro al merito civile, di cui Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono stati insigniti, testimoniano il valore che la Repubblica riconosce al loro sacrificio e sono anche un'occasione per non dimenticare quanto la libertà di stampa rappresenti un presupposto fondamentale per lo Stato di diritto.

dolore che in un giorno primaverile, dove l'anima si predispone al futuro, al bello, al rilassamento, ai semi che diventano piante più o meno importanti, parlare della morte

Così come quando domani parleremo di infortuni sul lavoro, cosa è più distonico di morire o di ferirsi per sempre per lavorare, il primo diritto della Costituzione. Ilaria, pur essendo una persona rasserenante e in qualche modo rasserenata, cercava di descrivere l'inferno, i dolori organizzati, i dolori singoli, con una forza di analisi, ma anche di coraggio,

manifestavo la mia preoccupazione sul traffico dei bambini, tanto che dissi, in quel periodo così particolare della mia vita, per la delinquenza organizzata internazionale un chilo di bambino vale come un chilo di eroina. fu attenta non tanto perché lo dicevo io, ma per l'argomento e anche per questo ha messo a repentaglio e - ahimè - ha addirittura pagato con la vita la sua necessità di far luce. Noi non lo abbiamo fatto in trent'anni con depistaggi, false informazioni, false dichiarazioni. C'è voluta la bravura della giornalista Cazzaniga per dire che il testimone contro Ilaria era un falso. Voglio dire questo, Presidente, colleghe e colleghi: a che serve commemorare? Serve certamente a rinnovellare la memoria e questo è utile - ma soprattutto a dare nuovo impulso alla voglia di far chiarezza. È vero che nel nostro Paese così meraviglioso e fortunato, in parte, tante cose oscure devono ancora venire alla luce, ma cominciamo da un punto, quello di Ilaria. Lo dobbiamo a lei, al suo operatore, ai genitori, a chi l'amava, a chi l'ama ancora. Un nuovo impulso per portare luce dove non c'è la luce, Presidente, fa sempre bene e non abbaglia mai l'anima.

come lei ha rammentato, siamo oggi chiamati a ricordare - nel senso etimologico del termine, a rimetterci nel cuore le figure di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, che trent'anni fa hanno perso la vita in una vicenda drammatica e ancora non compresa fino in fondo. Ma, se non vogliamo apparire - come dicevano le Scritture, come i cembali che suonano a vuoto - non dobbiamo circoscrivere il momento della commemorazione all'interno di una retorica di circostanza. La drammatica vicenda di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ci interpella tutti e questi trent'anni non fanno che aumentare il peso di queste domande inevase, alle quali siamo pur tenuti a fornire alcune risposte. Questa storia ci porta a chiederci che Paese siamo, se dopo trent'anni non sappiamo rendere giustizia ai migliori di noi che si sono sacrificati. E ci interpella su che classi dirigenti siamo, se non riusciamo a costruire un sistema istituzionale, diplomatico, giudiziario che sia davvero in grado di dare le risposte a questo genere di domande, a questo tipo di interrogativi. Più in generale, signor Presidente, la vicenda di Ilaria Alpi ci interpella e ci pone un'altra domanda: che destino ci appartiene come Paese, se ogni morte sacrificale dall'inizio della storia di questa Repubblica, da Portella della Ginestra, andando avanti al caso Mattei, a piazza della Loggia, alla vicenda Moro fino a Ilaria Alpi, a Ilaria Alpi, porta con sé uno strascico inquieto e inevaso di risposte mancanti? Non che attorno a questa vicenda siano mancati gli strumenti, anzi inchieste, indagini e approfondimenti internazionali, addirittura Commissioni parlamentari, forse anche in qualche caso interpretate in maniera un po' particolare; ma certamente ci sono stati presunti tentativi di depistaggio, incarcerazioni, assoluzioni, richieste di archiviazione attorno a una vicenda che toccava situazioni molto complesse - come il Presidente ha ricordato - che le cronache ci consegnano. al lavoro coraggioso di una *reporter* vera, che creava e che credeva nelle condizioni di una libera informazione di un servizio pubblico e che quindi ci voleva raccontare cosa ci fosse in quella Somalia tormentata di tre decadi fa attorno ai temi del traffico delle armi e dello smaltimento illegale di rifiuti tossici. Tutta questa vicenda ci consegna anche un quadro inquieto che deve tenere aperta la nostra coscienza. Se vogliamo davvero fare in modo che questa sia non una commemorazione retorica, ma un elemento che ci consenta di poter portare il nostro contributo al disvelamento della verità, ci deve consegnare questo elemento di irrequietudine per non essere stati *pro quota* in grado di assicurare verità e giustizia fino in fondo. Attorno Attorno a questa vicenda possiamo davvero riscoprire le parole di quel poeta a cui si ispirò anche Hemingway in uno dei pezzi più belli della letteratura del Novecento - parlo della poesia di John Donne - quando ci diceva che non dobbiamo mai chiederci per chi suona la campana, perché la campana suona sempre per noi.

giornalista, fotoreporter del TG3, assassinata a Mogadiscio insieme al suo operatore Miran Hrovatin. Da allora, processi, Commissioni parlamentari e inchieste giornalistiche non sono riusciti a dare una soluzione e una risposta a questa tragedia. Ilaria giunse in Somalia nel 1992 per seguire, come inviata del TG3, una missione di pace promossa dalle Nazioni Unite, guarda caso per porre fine alla guerra civile che era scoppiata nel 1991 dopo la caduta di Siad Barre. Quando è stata uccisa, Ilaria stava seguendo in particolare il ritiro delle truppe statunitensi, che in quei giorni stavano lasciando il Paese. Prima arrivare lì, Ilaria era una giornalista che aveva studiato molto, aveva imparato la lingua, l'arabo; era stata

che stava investigando su un traffico di armi e di rifiuti tossici che avrebbe visto, tra l'altro, la complicità dei servizi segreti italiani e di altre istituzioni sempre italiane. di un traffico di rifiuti che i Paesi industrializzati dislocano molto spesso nei Paesi africani in cambio di tangenti e armi ai gruppi politici locali. Per ricordare e non far finta di niente, a distanza di trent'anni siamo ancora qui a ricordare l'abnegazione e la professionalità di Ilaria Alpi, la sua dedizione al lavoro che l'ha portata alla morte. Bisogna morte. Bisogna dirlo: Ilaria Alpi era una giornalista d'inchiesta non asservita ai potenti; era una persona che aveva la schiena dritta e che nessuno poteva condizionare: una lavoratrice ammazzata proprio perché

Il mondo occidentale, il mondo del benessere, il nostro mondo si deve domandare perché nel Continente africano scoppiano certe guerre. Quale

«C'è un filo invisibile che lega la morte di mia figlia alle navi dei veleni, ai rifiuti tossici partiti dall'Italia e arrivati in Somalia. Ci sono documenti che lo provano. Ci sono testimonianze dei pentiti. Eppure nessuno ha avuto il coraggio di processare i colpevoli.

Ci sono crimini che non hanno scadenza ed è preciso compito dello Stato accertare le responsabilità. Oggi c'è un'inchiesta giudiziaria formalmente ancora aperta alla procura di Roma. Mi auguro che si faccia luce cui finora ci sono stati depistaggi e capri espiatori e che si giunga ai veri responsabili e li si condanni, come meritano la memoria di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

con una raffica di kalashnikov poco lontano dall'ambasciata italiana di Mogadiscio, in Somalia. La giornalista e il cineoperatore erano lì per seguire, per conto del TG3, il ritiro delle truppe statunitensi dal Paese, dove era in corso da anni una guerra civile. I due stavano parallelamente indagando anche su un traffico internazionale di armi e di rifiuti tossici che, secondo alcuni, avrebbe coinvolto anche società italiane legate forse alla cooperazione internazionale. Nonostante le indagini in questi anni si siano moltiplicate, tra inchieste giudiziarie e una Commissione parlamentare votata dal Parlamento nel 2004, dopo incarcerazioni, assoluzioni e richieste di archiviazione, purtroppo la verità non è ancora venuta a galla e non sono stati individuati né gli esecutori né i mandanti.

il cittadino somalo che è stato accusato anche da altri due testimoni: Sid Abdi, autista di Alpi e Hrovatin, e il testimone oculare Ali Ahmed Ragi. de «La Stampa» l'ambasciatore nega il depistaggio e che le accuse nei suoi confronti sono prive di ogni riscontro, ma le dichiarazioni del nuovo testimone meritano comunque un attento vaglio da parte dell'autorità giudiziaria. La vicenda è assai intricata ed opaca.

dopo che una *troupe* della trasmissione «Chi l'ha visto?» riuscì a intervistare il testimone Ragi, che raccontò di aver falsamente accusato Hashi *Assan* in cambio di un visto per lasciare la Somalia. Quest'ultimo, Hashi Assan - è un ulteriore particolare assai inquietante - è morto saltando in aria al suo rientro in Somalia nel 2022, dopo aver peraltro ottenuto un risarcimento cospicuo da parte dello Stato italiano per l'ingiusta detenzione subita. Nonostante il tempo passato renda sempre più difficile trovare riscontri obiettivi, la ricerca della verità deve proseguire, in memoria delle vittime e per rispetto del loro lavoro e della loro testimonianza. A sua volta, la procura della Repubblica di Roma deve proseguire le indagini, che peraltro non si sono mai concluse, interrogando - credo al più presto - un nuovo testimone, intervistato oggi su «La Stampa». In questo tragico anniversario, quindi, signor Presidente, Forza Italia si vuole stringere ai familiari e ai colleghi di Ilaria Alpi e *Miran* Hrovatin, al TG3 e alla sua redazione, con la speranza che gli assassini e i mandanti siano finalmente assicurati alla giustizia. *(Applausi)*.

e Miran Hrovatin molti sono i ricordi che affiorano alla mente. Era il dicembre del 1993 e io terminavo la mia missione da casco blu dell'ONU in Somalia. Somalia. In quel periodo percorrevo le stesse strade di Ilaria e Miran di Mogadiscio; solo che io di lì a breve, dopo quattro mesi di servizio che avevo prestato ai confini con l'Etiopia, sarei ritornato in Italia, mentre Ilaria e Miran iniziavano quella loro indagine giornalistica che di lì a breve li avrebbe portati alla morte,

Oggi, dopo trent'anni, possiamo affermare che l'omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin rientra a pieno titolo nei casi più bui e misteriosi della nostra Repubblica. Nessuno è stato mai condannato in via definitiva per questi omicidi. L'unico ad essere stato inizialmente condannato e incarcerato fu il cittadino somalo Hashi Omar Hassan, che successivamente, dopo diciassette anni di reclusione, fu poi assolto per non aver commesso il fatto. Questo caso rimane avvolto nel mistero, con molte ipotesi che hanno confuso le acque e reso difficile stabilire la verità. Molte sono state le piste che si sono inseguite e portate avanti per l'omicidio, da un tentativo di rapimento per il riscatto finito male, a una vendetta contro ipotetiche violenze sui cittadini somali, di cui furono accusati i militari italiani in Somalia, o il presunto traffico illecito di rifiuti e armi tra l'Italia e la Somalia negli anni precedenti. Di sicuro, però, Ilaria Alpi con la sua inchiesta voleva mettere in chiaro quanto di oscuro ci fosse stato nel tempo e nei rapporti tra i due Stati, inchiesta che le è costata la vita. Negli anni sono stati dedicati degli omaggi a Ilaria Alpi, tra cui strade, giardini ed edifici. Per lei è stata creata una rosa, di cui un'esemplare cresce nella sede della Rai. Dal 1995 a Riccione il premio Ilaria Alpi viene assegnato alle migliori inchieste televisive italiane dedicate ai temi della pace e della solidarietà: occasioni sicuramente lodevoli per ricordare il suo coraggio e il suo impegno. Tuttavia, però, non basteranno fino a quando non si arriverà alla verità e non ci sarà giustizia. Fino al 2014 la madre di Ilaria, Luciana Ricciardi, chiedeva ai vertici di chiudere il premio giornalistico, perché giustizia non era stata fatta sulla morte della figlia. I genitori di Ilaria sono morti senza conoscere la verità sulla morte della figlia. È arrivato, Presidente, dopo trent'anni, il momento di dare un nome ad assassini e mandanti. Il nostro Capo dello Stato si è unito alla richiesta di ricostruire i fatti di quel 20 marzo. Gli assassini e i mandanti sono ancora senza nome e senza volto, dopo indagini, depistaggi, ritrattazioni, processi finiti nel nulla. È una ferita che riguarda l'intera società. Le istituzioni sanno che non ci si può mai arrendere nella ricerca della verità. Il messaggio del nostro Presidente si è concluso con un monito contro le limitazioni alla libertà di stampa. Il valore dell'autonomia della stampa libera è sotto attacco in tante parti del mondo. Molti giornalisti pagano con la vita la loro indipendenza dai poteri, la loro ricerca di verità. Il ricordo di Alpi e Hrovatin suona da impegno a rimuovere gli ostacoli alla libertà di informazione, ovunque si manifestino. Mi conceda, Presidente, di rivolgere un pensiero anche a tutti i militari e civili italiani che hanno dato la loro vita o sono rimasti feriti, prestando servizio nella missione umanitaria

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: due nomi che siamo abituati ad ascoltare uniti. Ne parlano i telegiornali e i giornali da trent'anni, perché uniti hanno lavorato, uniti hanno trovato la morte e unico è stato il loro destino, in quanto ancora oggi non si sa che cosa davvero sia accaduto, né chi sia stato davvero ad ucciderli, né chi siano stati - soprattutto direi - i mandanti. Ilaria Alpi quando è morta, trent'anni fa, aveva anni. Per me era un'adulta; io ne avevo sedici e vedevo il suo bellissimo volto al telegiornale. Non capivo esattamente di cosa stessero parlando e ancora oggi in tanti non hanno voluto che capissimo di cosa si stava parlando. Era una donna che aveva fatto tutto quello che poteva fin da piccola per intraprendere la carriera di giornalista d'inchiesta. Fin dalla scuola scriveva sul giornalino scolastico, aveva avuto una borsa di studio per entrare in Rai. Parlava l'inglese, il francese e anche l'arabo perché, per un giornalista d'inchiesta, è molto importante conoscere la lingua, possibilmente la lingua che viene parlata sul posto. È stata in Somalia per la guerra civile, e ci è tornata per scoprire che cosa stesse succedendo. Ricordo che erano anche gli anni

sul traffico illecito di rifiuti tossici in cambio di armi. Si trattava di un Paese in via di sviluppo per cui si era fatto tanto o meglio si era cercato e si era detto che si sarebbe fatto tanto per la cooperazione e per l'aiuto umanitario.

Pensate che cosa potesse provare lei, forse anche un sentimento di schifo perché è questo che rappresenta bene la situazione, di fronte ad una popolazione che usciva da una guerra civile, che stavamo cercando di aiutare, usata per scopi economici, senza alcun ritegno, senza nessuna coscienza e senza alcuna morale. Lei e Miran hanno cercato di scoprire la verità. Non erano al soldo dei potenti, come spesso accade per i giornalisti d'inchiesta e come spesso accade per i giornalisti d'inchiesta che vengono ammazzati, e insieme hanno trovato la morte. stata aperta un'indagine dalla procura di Roma per Ilaria Alpi e a Trieste per Miran. Ancora oggi c'è un fascicolo aperto presso la procura di Roma, ma nel frattempo i genitori di Ilaria sono morti senza conoscere la verità. Sappiamo che qualcuno è stato sedici anni in galera da innocente e, quando finalmente è stato dichiarato innocente, è stato ammazzato. Quindi mi pare abbastanza evidente - non a me, ma dagli dagli atti delle indagini - che ci sia qualcosa di davvero molto grave dietro queste morti. La morte di Ilaria, che noi vogliamo ricordare insieme a quella di Miran oggi, è la morte di troppi giornalisti di inchiesta, che mettono l'anima nel lavoro che fanno. È un giornalismo diverso da quello comune, senza nulla togliere a chi fa questo mestiere, ma è molto, molto più pericoloso. Sono 1.600 i giornalisti uccisi nell'ultimo trentennio e sono 400 quelli ad oggi ancora incarcerati. La mamma di Ilaria diceva una cosa molto importante: non cerco giustizia, voglio solo conoscere la verità. La verità che cercava Ilaria è la verità che noi oggi abbiamo il dovere di cercare per lei e per tutte le persone che sono morte senza una spiegazione. Questa è un'inchiesta che Ilaria sicuramente avrebbe voluto fare, magari proprio insieme a Miran Hrovatin.

per fare il loro mestiere, in una zona di guerra, di carestia, di guerra civile, dove né la missione ONU Restore Hope né quella italiana Ibis avevano saputo portare

avevano così scoperto che, all'ombra della cooperazione internazionale, si svolgevano degli illeciti e traffici coperti di armi e rifiuti speciali. vennero ammazzati per questo. Per tanti anni, i genitori di Ilaria, Luciana e Giorgio, che oggi non ci sono più, hanno dedicato il loro strazio e la loro ferita non rimarginabile a cercare la verità. Era commovente entrare nel loro soggiorno e vedere la foto di Ilaria sorridente, come se fosse ancora lì. Nella ricerca della verità trovavano una ragione di vita. di una verità mai trovata, perché ostacolata da errori, depistaggi, omissioni e forse superficialità nelle prime indagini. In questo impegno, Luciana e Giorgio Alpi sono stati sostenuti da settori della politica e dai colleghi del TG3. Indimenticabile la commozione di Flavio Fusi, suo collega, quando dovette annunciare in diretta, al suo telegiornale, la notizia

io credo sia giusto ricordare come costante nel tempo sia stato il sostegno della Federazione della stampa, dell'ordine dei giornalisti, di associazioni come Articolo21, Liberainformazione e del comitato "Noi non archiviamo", di cui portavoce è Mariangela Grainer, una ex parlamentare. Altri giornalisti, ancora oggi, ancora in queste ore - come ricordava il senatore Zanettin - scavano,

di Ilaria, Federica Sciarelli, che insieme a Chiara Cazzaniga, inviata di «Chi l'ha visto?», ha saputo dare una svolta alla vicenda. Chiara Cazzaniga scoprì, non lontano da Londra, uno dei primissimi depistatori, Ahmed Ali Rage, soprannominato Jelle. Questi le rivelò di avere mentito su indicazione di italiani, non meglio precisati, accusando dell'omicidio *Hashi* Omar Hassan,

Luciana e Giorgio Alpi andavano a trovarlo, perché lo sapevano innocente. Grazie all'inchiesta di Cazzaniga, si riuscì a fare la revisione del processo e Hashi venne scagionato e liberato. Eravamo anche noi, quel giorno, presso la corte d'appello di Perugia e io ricordo, quando venne pronunciata la sentenza di definitivo proscioglimento, come Luciana Alpi abbracciò quell'omone, *Hashi* Omar Hassan, che sapeva innocente. Egli tornò in Somalia libero, ma dopo poco tempo venne assassinato con una bomba piazzata nella sua auto. Per tale ragione, in questo trentesimo anniversario, le parole verità e giustizia non debbono suonare retoriche. Noi abbiamo interpellato il procuratore Lo Voi e andremo a conferire come Comitato con lui per portare elementi e fatti che motivano la necessità, come detto dal senatore Guidi, di un nuovo impulso alle indagini. Che altro deve succedere, dopo l'assassinio di Hashi con la bomba, per non riaprire queste indagini con grande determinazione? Ancora una volta è stato il presidente Mattarella a trovare le parole giuste in questo anniversario, rendendo onore ai due giornalisti, parlando di ignobili traffici, depistaggi e dicendo una frase chiave: le istituzioni sanno che non ci si può mai arrendere nella ricerca della verità e nel rimuovere gli ostacoli alla libertà di informazione. È importante che concetti simili li abbiano espressi anche i Presidenti delle Camere e la stessa Presidente del Consiglio. Ora noi chiediamo che queste parole vengano sempre tenute presenti e si trasformino in

a grandissima maggioranza, ha votato un atto molto importante, lo European media freedom act, che rappresenta un atto forte e da applicare a difesa della libertà di informazione, del giornalismo di inchiesta e del servizio pubblico, quello per cui sono morti Ilaria e Miran e altri giornalisti. Mi piace citare delle donne coraggiose: Maria Grazia Cutuli, Daphne Caruana Galizia, Anna Politkovskaja. Questo giornalismo costituisce ancora oggi un presidio fondamentale per una cosa che è sotto attacco e che si chiama democrazia. Questo impegno, nel trentesimo anniversario di quell'assassinio, deve essere coerente, coerente, deve essere il modo migliore per onorare la memoria di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

insieme al collega e cineoperatore triestino Miran Hrovatin. Era lì a Mogadiscio, come hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduta, come inviata del TG3. Era a fare il suo lavoro. Il lavoro che amava. La mamma Luciana, prima di andarsene per sempre all'età di ottantacinque anni, aveva ricercato la verità per ventiquattro anni, giorno e notte, instancabile, ma non è mai riuscita ad arrivare ad una verità. Il papà Giorgio, che chiedeva giustizia e verità, non ha mai saputo perché gli avevano portato via sua figlia in un modo così brutale. La verità è quella che cercano e poi raccontano i giornalisti. Il mio grazie va a tanti giornalisti che si battono per la verità. Siamo al loro fianco contro ogni forma di censura e imposizione del pensiero unico. Vorrei ringraziare tutti quei giornalisti che dai luoghi di guerra, assieme ai *reporter* e ai *fotoreporter*, rischiando la vita, ci raccontano quello che sta avvenendo in quei posti. Sono tanti quelli che, per garantire il diritto all'informazione e alla libertà, hanno dato e stanno dando la vita. A loro va il nostro ringraziamento. Parlavamo di verità, ma su Ilaria e Miran gli assassini e i mandanti sono ancora senza nome e senza cognome, senza volto, dopo indagini, depistaggi, ritrattazioni, processi finiti nel niente. È una ferita che riguarda l'intera società, l'Italia, la nostra Nazione. Oggi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato alla Camera Ilaria e Miran e ha ribadito a tutti noi l'impegno rispetto alla ricerca della verità. Parlando di Ilaria ha ricordato il suo coraggio. Il coraggio di una donna che non le ha permesso però di riabbracciare i suoi cari. Per noi Ilaria è un esempio. Una cosa è certa: non ci arrenderemo nella ricerca di verità, continueremo a cercarla, è un nostro dovere. Faremo di tutto affinché anche questo non rimanga uno dei misteri della nostra Nazione, nel segno di Ilaria.

dei trasferimenti di queste Olimpiadi, che come sappiamo sono delocalizzate su diverse località e quindi pareva utile creare un piano e una programmazione in modo che si coordinasse la mobilità su tutto il territorio interessato, da Milano a Cortina, da Verona a Bormio. Un piano eviterebbe di trovarsi nelle circostanze contestuali in difficoltà per mancata coordinazione.

come tutti sappiamo oramai, i due canoni di riferimento di questi Giochi olimpici sono la sostenibilità economica e quella ambientale.

valorizzare economicamente i sacrifici dei servizi ecosistemici o, viceversa, il guadagno degli stessi. Tutto ciò semplicemente per trasparenza, per mettere nero su bianco l'eventuale successo dell'organizzazione di questa manifestazione. L'emendamento non è stato accolto e immagino che forse questa sostenibilità ambientale non sia proprio rispettata.

ricorrendone le esigenze, di dare soluzione ad eventuali questioni che potrebbero sorgere al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026 in relazione al regime proprietario delle opere necessarie allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici e paralimpici».

Signor Presidente, vorrei fare un breve intervento su questo emendamento della collega Sironi per dichiarare il nostro voto di astensione e per dire che, per quanto ci riguarda, le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 rappresentano una importante occasione dal punto di vista economico, turistico e sportivo per tutto il nostro Paese. Avremmo però voluto che ci fosse un approccio culturale diverso da parte del Governo e di tutte le istituzioni interessate. Avremmo voluto che questo evento si declinasse in un modo più sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, in un territorio in cui il consumo del suolo e i cambiamenti climatici hanno già mostrato diversi effetti collaterali. È per questa ragione che avevamo fatto altre proposte: ad esempio, avevamo detto che il villaggio olimpico di Cortina non si realizzasse dove aveva previsto il Governo, ma si realizzasse recuperando il villaggio di Borca di Cadore, sede

Con l'emendamento della collega Sironi sono alla nostra attenzione tutti i problemi e le criticità relative alla pista da bob. A tale proposito, vorrei che l'Assemblea sapesse che, per quel che riguarda questo impianto, se tra un anno e cioè a marzo 2025 l'impianto non supererà il test di preomologazione, scatterà il piano B richiesto dal Comitato internazionale olimpico, come peraltro confermato da un recente sopralluogo avvenuto in Veneto qualche settimana fa. Il piano B è la trasferta all'estero. Tutti conosciamo le lungaggini, i balbettii, le inadeguatezze e l'incertezza che c'è stato su questo progetto da parte della Regione Veneto e da parte del Governo. Sappiamo dei bandi andati deserti e delle legittime preoccupazioni che sono state avanzate sull'impatto ambientale. Sappiamo anche delle opinioni diverse che ci sono all'interno del Governo e che si sono manifestate. Ciò che dobbiamo evitare, però, è che il nostro Paese faccia una figuraccia dal punto di vista internazionale. Siccome vogliamo ancora una volta ricordare, per esempio (perché qui parliamo di infrastrutture) che che la variante di Cortina non si realizzerà per il 2026, sarebbe bene che il Governo dicesse qualcosa in proposito,

dopo l'ultimo bando che è avvenuto, è assolutamente necessario prevedere tutte le risorse economiche per ripristinare dal punto di vista naturale quell'opera e le risorse economiche per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria di quell'impianto che non possono essere affidate ovviamente solo alle istituzioni locali e al Comune di Cortina. è che questi Giochi sono una grande opportunità, ma dovevano essere a costo zero, con un'importante *legacy* che invece non si sta realizzando e piuttosto con un costo altissimo in termini economici ed ambientali. Accanto a questo ribadiamo che quelle opere stradali che dovevano essere realizzate non verranno realizzate. È vero che in questo decreto-legge non si parla della pista da bob, ma è altrettanto vero che noi abbiamo voluto porre il tema alla vostra attenzione e continueremo a farlo con tutti gli strumenti parlamentari a disposizione, ritenendo questa una sfida importantissima che deve rappresentare, però, una chiave diversa per una realtà sostenibile dal punto di vista economico e sociale.

sulla dichiarazione di voto del collega. In realtà tutte le sue argomentazioni sembravano portare ad un voto favorevole, piuttosto che ad un'astensione. Con questo emendamento richiamo in particolare ciò che riguarda le spese di gestione e manutenzione dell'impianto, che non possono essere accollate agli enti locali.

Il Movimento chiede che per la realizzazione delle opere complementari connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, si tenga conto per ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere dell'indicatore dell'impronta di carbonio per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN

che venissero misurate attraverso questi indicatori le variazioni di tali fattori, anche nell'ottica di una gestione del territorio e di un'eventuale pianificazione futura. Non ho ancora ascoltato il parere del Governo e del relatore

che ha una certa complessità. Questo emendamento, infatti, è volto a potenziare la struttura dell'autorità di bacino, in particolare l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali.

Lo spunto di questo emendamento è un invito al Governo a fare una considerazione su certe normative, che sono veramente molto burocratiche e a volte vanno ad appesantire i percorsi per l'adozione del piano di assetto del territorio, del piano degli interventi,

anche per accelerare l'esecuzione di alcuni lavori. Dobbiamo veramente fare un ragionamento, in Italia, su quella che è la nostra capacità strutturale, dal punto di vista ordinamentale, normativo, ma anche di progettualità all'interno degli enti locali. di poter adottare i progetti, realizzare le opere, spendere anche i denari che noi stanziamo. C'è infatti un serio problema in Italia, come si è visto anche con l'adozione del PNRR.

Grazie, Presidente. nella direzione auspicata. È un passettino verso la consapevolezza della necessità di monitorare e pianificare attentamente fenomeni di dissesto idrogeologico. È quindi un passettino che merita la nostra astensione.

Signor Presidente, presto volentieri la voce alla collega senatrice Versace. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi... chiedo ai colleghi di uscire dall'Aula mantenendo per favore un minimo di silenzio in modo che possiamo ascoltare tutti la dichiarazione di voto. LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Grazie, Presidente. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e della *governance* della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 SpA. In sintesi il testo individua nell'ANAS SpA il soggetto che dovrà attuare le opere complementari in ambito stradale e interviene anche sulla struttura gestionale della società Infrastrutture Milano Cortina, con particolare attenzione alle funzioni attribuite ai membri dell'organo di amministrazione. In particolare si prevede, all'articolo 2, che i componenti dell'organo di amministrazione del collegio sindacale siano designati e non nominati, passando così da un sistema di nomine da parte delle amministrazioni centrali e regionali a un modello in cui la nomina è affidata all'assemblea dei soci, responsabilizzando gli azionisti nella scelta degli organi sociali. Partendo dunque da quella che sarà la struttura della nuova compagine societaria e quindi della responsabilità ad essere riconosciuto, vorrei ringraziare l'8a Commissione del Senato referente sul provvedimento per aver accolto le proposte, appunto, degli emendamenti presentati dalla mia collega senatrice Giusy Versace, che sono a noi molto cari, in particolare su alcuni punti. Il primo è riferito alla *governance* della società in considerazione del fatto che gli eventi richiedono la realizzazione del completamento straordinario e urgente di azioni e interventi relativi anche alla mobilità e all'accessibilità. In particolare, nel testo originario dell'articolo 2, erano chiamati a designare tre componenti dell'organo di amministrazione della società: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'autorità di Governo competente in materia di sport. Ora, con l'emendamento proposto dalla collega Versace e accolto dai componenti della Commissione, si prevede il coinvolgimento anche dell'autorità di Governo competente in materia di disabilità nella designazione del consiglio di amministrazione del collegio sindacale e che dovrà essere garantita una maggiore attenzione alle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità. Signor Presidente, per noi il tema della disabilità e dell'accessibilità è fondamentale in quest'opera.

e non invece su Bormio Valdisotto, perché queste sarebbero occasioni per rendere accessibili le strutture non solo per gli atleti paraolimpici, ma anche per le persone con disabilità e per i loro familiari. Dovremmo cogliere queste occasioni, che sono importanti per il Paese, per farci compiere un passo in avanti non solo per gli eventi - in questo caso molto importanti - ma anche per ciò che succederà dopo

la corsa a ostacoli, anzi - se mi consente, visto il tema dei giochi invernali - lo *slalom* speciale che ci troveremo ad affrontare, porterà all'avvio e alla chiusura dei cantieri prima dei termini consigliati. Ma c'è un punto

Ci dobbiamo porre il tema della sostenibilità economica di queste opere dopo le gare olimpiche, perché abbiamo già avuto altri esempi di forti investimenti forti investimenti pubblici nella realizzazione di questi grandi eventi che però, se non hanno le coperture in materia di manutenzione degli impianti, rischiano poi di creare dei disavanzi di bilancio. In questa discussione abbiamo sentito molto evocare il tema della sostenibilità ambientale, un tema sicuramente importante, ma non abbiamo sentito parlare con altrettanta chiarezza del tema della sostenibilità economica e finanziaria. Questo è il tema della *legacy*: cosa rimarrà della manutenzione di questi impianti dopo i grandi eventi? Il rischio che questi costi ricadano sulle amministrazioni comunali, e che quindi sarà difficile

perse, gettate via, per la crescita di interi territori e non solamente di Roma, come è avvenuto pochi anni fa, ci apprestiamo a cogliere un'occasione fondamentale e importante discutendo questo decreto-legge che ridefinisce gli interventi in vista in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Siamo consapevoli che se vogliamo vincere questa sfida dobbiamo farci trovare pronti a combatterla bene, per vincere effettivamente la sfida che si porrà come cartolina dell'Italia agli occhi del mondo. Infatti le Olimpiadi,

inoltre, rappresentano un momento imprescindibile di sviluppo economico ed infrastrutturale: oggi le Olimpiadi rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi, sono il simbolo della pace e della fratellanza fra i popoli che si riuniscono nel nome dello sport e si confrontano in modo leale. L'ideale olimpico viene espresso attraverso la stessa bandiera, i cinque cerchi di colore diverso che rappresentano i continenti e si sovrappongono parzialmente in un abbraccio ideale; un simbolo che, alla luce di quanto accade nel mondo in questo periodo, assume un significato ancora più importante. L'Italia ha ospitato i giochi in tre occasioni: le Olimpiadi invernali a Cortina d'Ampezzo nel 1956, i Giochi olimpici qui a Roma nel 1960 e i Giochi olimpici invernali nel 2006 a Torino.

Già da tempo sono in corso progetti per costruire i nuovi impianti, i villaggi per gli atleti, i collegamenti con le piste. È un'occasione che non possiamo mancare. I Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano, dunque, una grandissima opportunità per le Regioni coinvolte, Lombardia e Veneto, e per tutta l'Italia perché, quando ci sono eventi così importanti, l'indotto si riflette positivamente su tutto il Paese. Vogliamo farci trovare pronti e sono certo che faremo le olimpiadi migliori, anche attraverso strumenti normativi come il presente decreto-legge, che auspico possa trovare la maggiore convergenza di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Il Governo Meloni, i Ministeri competenti e le amministrazioni regionali e locali stanno lavorando alacremente per questo obiettivo. Siamo consapevoli che tanto è stato fatto e tanto ancora c'è da fare. Secondo autorevoli fonti, i Giochi olimpici invernali avranno un impatto sul PIL di 3 miliardi, con un investimento previsto di circa un miliardo. Inoltre, l'evento dovrebbe produrre un incremento di risorse all'interno del singolo comparto dello sport pari a un miliardo e 142 milioni di euro, mentre gli altri settori beneficeranno di maggiori risorse per un miliardo e 26 milioni. In altri termini, un aumento di domanda di un miliardo nel comparto dello sport genererà un effetto positivo su tutto quanto il settore economico nazionale di circa 3 miliardi. L'organizzazione delle Olimpiadi invernali sarà quindi un volano sia da un punto di vista occupazionale, sia da quello della produzione per le imprese fornitrici del comparto sportivo. Si prevede una crescita dell'occupazione di circa 13.000 unità,

Non possiamo dimenticare che i flussi turistici in arrivo in occasione della *kermesse* olimpica non saranno brevi. Si prevede quindi che oltre il 60 dei visitatori avrà una sosta di tre-sette giorni e questo farà sì che potranno avere un beneficio non solamente le zone limitrofe a quelle dove saranno gli eventi ma anche il resto d'Italia, per conoscere la patria della qualità e della bellezza, andando a sostenere così il turismo enogastronomico, culturale, monumentale e paesaggistico dello splendore che riveste l'Italia in tutte le sue parti. Questa grande avventura è iniziata con la certezza che le Olimpiadi del 2026 possano simboleggiare il domani, la ripresa e un'occasione di sviluppo economico: si creeranno posti di lavoro oltre a quelli già registrati

Esse fanno parte del domani che va costruito oggi ripartendo dallo sport, come abbiamo dimostrato, grazie anche a un decreto-legge che ha la sua urgenza nella necessità di attuare delle opere connesse alle opere complementari, proprio come è stato fatto la settimana scorsa con il decreto-legge per il G7 in Puglia. Al fine di accelerare e di garantire, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi nelle Olimpiadi invernali nel 2026 nella Regione Lombardia, nella Regione Veneto, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attività turistica, dei citati territori, è stata autorizzata una specifica *governance*. La revisione di quest'ultima muove dall'esigenza di distinguere i compiti tra i diversi membri dell'organo di amministrazione, al fine di assicurare una efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità, anche in considerazione delle attribuzioni commissariali su opere connesse e non affidate ad ANAS.

Approviamo questo decreto-legge lavorando insieme, al di là dei campanilismi e delle differenze politiche, affinché queste siano ricordate come le migliori Olimpiadi, non solamente a livello italiano.

è sempre stata a favore dello sport, dei piccoli e grandi eventi sportivi, quindi come tale ha dato sempre grande attenzione a questo tema. Siamo stati in prima linea per inserire lo sport in Costituzione, così come abbiamo lavorato su tanti disegni di legge in materia. Anche in questa sede voglio ringraziare il Governo, che spesso ha accolto positivamente questo lavoro fatto assieme, proprio perché è uno di quei temi che non dovrebbero dividere il Parlamento. Tale premessa è necessaria per spiegare invece le ragioni che ci vedono su molte questioni ancora con

tutto, voglio ricordare che mancano 687 giorni all'inaugurazione dei Giochi olimpici invernali assegnati a Milano Cortina; mancano cioè meno di due anni a questa importante cerimonia di apertura che si svolgerà venerdì 6 febbraio 2026 allo stadio Meazza di Milano. Ne sono però passati quasi cinque da quel 24 giugno 2019 in cui avvenne l'assegnazione a Losanna.

ai 2,2 miliardi di euro stimati due anni fa, i costi complessivi continuano ad aumentare. ha messo intanto le opere in sicurezza, accollandosi anche la garanzia della copertura finanziaria. Sappiamo però anche quello che sta accadendo

Torino dopo le Olimpiadi ha cambiato volto, è diventata davvero un'altra realtà, una città turistica vera e propria, perché perché quegli investimenti hanno dato la possibilità - lì sì davvero, collega Salvitti - di diventare un volano per Torino, per il Piemonte e per tutta l'Italia. Qui rischiamo - io spero di no - di non avere le stesse opportunità, perché siamo veramente indietro e sono tutti soldi pubblici quelli che si stanno spendendo. Allora voglio capire perché sulla *governance* avete avete insistito così tanto per cambiare tutto, solo perché tutte le scelte appartenevano a un Governo precedente. Ma se quelle erano scelte giuste, perché non continuare su quella strada? No, perché ancora una volta qualcuno doveva metterci le mani e decidere diversamente, solo per propaganda elettorale. elettorale. L'impressione è che oggi, rispetto alle manifestazioni e alle aspettative organizzative, siamo indietro. Io, Presidente, vorrei ricordare le parole che appartengono a un collega di Governo del ministro Salvini, che è il ministro dell'economia Giorgetti, il quale qualche tempo fa ha detto a Milano: mi sono pentito di aver portato le Olimpiadi e vedo che ci sono delle grandi difficoltà nella realizzazione delle opere. Quando verrà attivato lo spirito imprenditoriale? Mancano poco meno di due anni. Quando realizzeremo queste opere infrastrutturali? Questo l'ha detto un Ministro della stessa parte politica della Lega, in questo caso, e del ministro Salvini. Le nostre preoccupazioni sono proprio queste: ce la faremo a realizzare queste opere nei tempi previsti? La pista della discordia da bob a Cortina è in costruzione, dopo uno scontro politico nella maggioranza. La ditta Pizzarotti si è impegnata a consegnare la pista entro marzo 2025, cioè fra circa un anno, olimpico internazionale e dalla Federazione internazionale. Ma perché, per esempio, come ha detto la collega Fregolent stamattina, non utilizzare una pista già esistente e funzionante che è a Torino? Perché in questo modo si rischia, se quell'opera non sarà pronta (per pochi atleti, peraltro), di andare all'estero, di portare quella pista della discordia da un'altra parte, fuori dall'Italia. Allora, quale volano è per il nostro Paese? Quale opportunità produttiva e occupazionale? Questa pista costa già 120 milioni e comunque andrà conclusa, ma forse si arriverà dopo i Giochi. Per questo la Corte dei conti del Veneto ci vuole vedere chiaro e ha posto la propria attenzione proprio sull'organizzazione, con i costi così elevati, che continuano ad aumentare anche con incarichi pagati in maniera molto importante. I magistrati contabili hanno messo nel mirino la costruzione delle infrastrutture, compresa la pista inclusa. La conferma è venuta dall'inaugurazione, pochi giorni fa, dell'anno giudiziario 2024 a Venezia, con le relazioni del procuratore regionale Montella e del presidente della sezione di controllo Locci. La Corte dei conti evidenzia che rimangono «inalterate «inalterate le perplessità e le osservazioni già evidenziate nella precedente relazione di parifica del 2022, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dalla Regione ai fini della semplificazione della *governance* delle Olimpiadi». Era stato già evidenziato il fatto che molti enti si occupavano dello stesso soggetto, con il rischio di generare sprechi e doppioni e ora il ministro Salvini alla ditta Simico, la società che gestisce i lavori per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano e Cortina, ha aggiunto anche l'ANAS. In questo modo sappiamo che oggi la società Simico è nel mirino della Corte dei conti per un preoccupante ritardo, non essendo presente un quadro che possa dirsi definito e certo delle opere indifferibili e urgenti da realizzare. Insomma, l'attenzione della Corte dei conti è molto chiara e si è concentrata anche sulle due varianti di Longarone e Cortina,

state già abbondantemente spese, e rispetto anche ai ritardi con cui è stato attivato il tessuto imprenditoriale ricchissimo del Nord-Est ma anche della Lombardia, è perché non c'è stato un lavoro, una valutazione precedente, quando è stato assegnato a Milano Cortina questo grande evento sportivo, cioè nel 2019. Si sono persi tutti questi anni perché si doveva cambiare la *governance*, si doveva ricominciare daccapo. daccapo. Noi ci auguriamo che nonostante tutte le difficoltà, nonostante anche l'occhio attento della magistratura, si possa oggi procedere celermente a dare quelle opere infrastrutturali a Milano, alla Lombardia e a Cortina in modo particolare, cercando di tutelarla anche dal punto di vista ambientale, perché le due cose non devono essere messe necessariamente in contrapposizione. Credo che un intervento politico lungimirante - mi avvio a concludere, Presidente - si faccia in maniera diversa e che questa sia una grande opportunità. Pensate a cosa è stata Roma senza le Olimpiadi, proprio per la mancanza di lungimiranza di una sindaca come Virginia Raggi del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*; una grande opportunità sprecata per la nostra capitale. Però, siccome parliamo di soldi pubblici, mettiamoci davvero la testa, mettiamoci attenzione. Per tutte queste ragioni, Presidente, per le ombre e le luci che ci sono in questa situazione, il Gruppo Italia Viva, il Centro-Renew Europe, darà voto Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti di Governo, se mi avessero chiesto un paio di anni fa come mi immaginavo le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, da modesta ex atleta di sport invernali, mi sarei immaginata l'organizzazione di questo evento all'insegna del rispetto della natura e della tutela del paesaggio, perché è questo che ci è stato insegnato quando ci si allenava sulle piste e quotidianamente eravamo a contatto con la natura e la montagna. Mi sarei aspettata entusiasmo, coinvolgimento dei territori e dei cittadini di fronte ad un simile spettacolo e mi sarei anche aspettata la promozione di un turismo alpino caratterizzato da una mobilità dolce, perché sappiamo benissimo - l'ha detto anche la collega che mi ha preceduto quanta fatica si fa ad accedere ai comprensori montani. Invece, quello che vedo quando si parla dei Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026 è malcontento e frustrazione della popolazione, devastazione che la costruzione di future carcasse sta portando nei territori di gara, luoghi di altissimo valore paesaggistico e naturalistico deturpati da una politica che sta trascurando di fatto il benessere dei territori e dei suoi cittadini. Ciò che sento, e sono sincera, è la tristezza e la malinconia trasmesse dal suono del violoncello di Mario Brunelli, come è già stato detto in sede discussione generale, che ha accompagnato a Cortina l'abbattimento dei larici storici: musica che si è opposta alle motoseghe che stanno facendo spazio alla nuova pista da bob. Ripeto, è un'opera inutile, controversa, che non vuole nessuno e che, sulla scia di un dannoso spirito nazionalistico, il ministro Salvini ha deciso di costruire in tempi *record*. Stando alle strette tempistiche di realizzazione, la pista da bob dovrà essere consegnata, a garanzia di sicurezza degli atleti, al più tardi tra un anno, nel marzo del 2025, per permettere loro di testarla adeguatamente. Sappiate che i lavori non sono ancora iniziati e il rischio che non venga ultimata è molto concreto. Ricordo anche che si impiegheranno 120 milioni di euro per realizzare questa pista da bob e che il comune di Cortina dovrà sostenere una spesa pari a circa un milione e 400.000 euro l'anno per la manutenzione e gestione dell'impianto. Questa mattina, in discussione generale, il collega Rosa ha riportato la disponibilità, da parte della Regione Veneto, di contribuire ai futuri costi di gestione della pista da bob. Voglio specificare, però, che nella delibera con cui la giunta della Regione Veneto si impegna a contribuire alla spesa non si indicano né le stime dei costi né le modalità di erogazione di questi fondi. Diciamo chiaramente che questi impegni e intenti, senza dati concreti, valgono come il due di picche. Il collega Rosa, che adesso non è in Aula, ha affermato che la pista da bob sarà l'unica, a livello mondiale, a ricevere il certificato Envision, che attesterà la sua sostenibilità. Innanzitutto, vorrei ricordare che queste sono valutazioni preliminari, fatte sul progetto di una pista da bob che non si è ancora cominciato a costruire; ad oggi manca un piano di sostenibilità futura. Pertanto, questa promessa di certificazione di un'opera ancora da realizzare francamente lascia il tempo che trova. È importante anche ricordare che, nel 2009, il comune di Cortina era stato costretto a chiudere la pista da bob originaria, la pista Eugenio Monti, in mancanza di solidi aiuti da parte della Regione Veneto e della Provincia di Belluno. Evidentemente la pista da bob non era stata considerata essenziale per il comparto turistico ed economico di Cortina. Pensate che sarebbero bastati solo 4 milioni di euro per farla ripartire.

e Innsbruck. La pista di Torino, purtroppo, non è funzionante. Così si è sprecato molto tempo, tanto da chiederci lecitamente se vedremo mai il completamento anche delle altre infrastrutture previste per le Olimpiadi, come anche delle stesse opere stradali, la cui realizzazione verrà affidata con il provvedimento oggi in discussione ad ANAS. È il caso della cosiddetta bretellina, così definita perché si usano tanto i diminutivi, lunga 650 metri, relativa al tratto stradale Cortina-Longarone; opera già prevista per i campionati mondiali di Cortina 2021, mai completata, poi reinserita nei progetti delle Olimpiadi 2026. Però, senza il completamento delle altre infrastrutture a cui è collegata, quali parcheggio e impianto di salita, ancora mai costruiti, essa sarà una lingua di cemento sospesa nel nulla. nel nulla. Oppure è il caso della tangenzialina di Bormio (un altro diminutivo): strada di 800 metri avente il costo di 7 milioni di euro, che verrà costruita nella golena di un torrente, in un'area ad alto rischio di dissesto idrologico. Così si stanno sprecando soldi pubblici, alle spalle dei cittadini, che nel caso dei Giochi olimpici, hanno visto lievitare il *budget* da un miliardo e 700 milioni a 4 miliardi. che si sta minando la credibilità e la reputazione del nostro Paese. Il decreto-legge che oggi siamo chiamati a votare è rappresentativo proprio di questo: il repentino cambio di *governance* di Simico, a due anni dalle Olimpiadi, e la delega ad ANAS sono la prova più evidente del fallimento della politica gestionale e organizzativa di questo Governo. Ricordo che a fronte della necessità di potenziare e ammodernare i trasporti ferroviari, a cui vengono destinati solo 400 milioni di euro, sono stati stanziati 3 miliardi per la costruzione di strade, senza contemplare l'impatto ambientale che il potenziamento del trasporto su gomma provocherà in termini di inquinamento atmosferico. Siamo stanchi di ribadire che già oggi ci sono 55.000 decessi annui per l'inquinamento atmosferico. non sono tanto sostenibili a livello ambientale, economico e sociale. Queste Olimpiadi ci avrebbero dato una grande possibilità di potenziamento delle linee ferroviarie ferroviarie ed è veramente frustrante sapere che l'Italia ha tutte le competenze e il *know-how* per procedere in questo senso e che è la classe politica al Governo il vero freno alla realizzazione di opere e infrastrutture sostenibili. Riprovevole infine è anche il fatto che non sia stata portata all'attenzione dei territori e delle comunità la realizzazione delle grandi opere previste per i Giochi. Non c'è stata un'interlocuzione politica con i cittadini; tutto è stato calato dall'alto a scatola chiusa. alle comunità montane e alle associazioni dei cittadini per l'immane lavoro che stanno facendo a tutela del loro e del nostro territorio. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra non siamo contrari alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, chiediamo solo che queste vengano organizzate e svolte nel modo più scrupoloso possibile e nel rispetto dell'ambiente, in modo da lasciare anche ai territori interessati un'eredità infrastrutturale futura che possa efficacemente essere utilizzata dalle comunità montane, già alle prese con i problemi legati allo spopolamento e alla scarsità di servizi; infrastrutture che incentivino al contempo un tipo di turismo responsabile e di qualità, che non gravi sulle risorse del territorio e che promuova con criterio le attività economiche connesse agli sport invernali, già gravemente in difficoltà a causa della mancanza di neve, che anche nel circo bianco questa stagione ha fatto cancellare ben venti gare di Coppa del mondo di sci. Spiace vedere che state traghettando questo Paese in tutt'altra direzione. Per queste ragioni, il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra esprime voto contrario a al provvedimento

straordinaria opportunità per promuovere il valore dello sport, l'importanza della sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica. Queste Olimpiadi sono un'opportunità imperdibile per rilanciare e valorizzare l'immagine dell'Italia nel mondo, la possibilità di mostrare le eccellenze italiane in diverse settori: dalla capacità organizzativa all'innovazione tecnologica, fino ad arrivare alla cultura e alla enogastronomia. Sarà un momento per dimostrare che l'Italia sa essere *leader* non soltanto nello sport, ma in molti ambiti, dando un messaggio di unità e di collaborazione internazionale. Milano e Cortina, come sedi di questo straordinario evento internazionale, garantiscono competenza nell'organizzazione di eventi di così grande portata. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si svolgeranno in un periodo storico caratterizzato da sfide globali senza precedenti, tra cui il cambiamento climatico, le tensioni geopolitiche e la difficoltà economica aggravata dagli esiti della pandemia e dalle guerre. Questo quadro ci pone davanti a diverse sfide significative per il futuro dell'evento. Penso alla sostenibilità ambientale; una delle principali sfide sarà quella di organizzare un evento che non solo limiti l'impatto ambientale, ma che contribuisca attivamente alla salvaguardia del pianeta. Ciò significa promuovere l'uso di energie rinnovabili, garantire che le infrastrutture siano sostenibili e che l'eredità degli impianti possa essere goduta anche dai nostri figli, dalle prossime generazioni. L'altra sfida è quella dell'innovazione della tecnologia; dovremmo essere in grado di sfruttare le ultime innovazioni tecnologiche per migliorare migliorare le prestazioni per gli atleti e per gli spettatori. Ciò significa organizzare un evento al passo con i tempi dal punto di vista digitale. Salute e sicurezza: dopo la pandemia, la salute e la sicurezza sono diventate ormai prioritarie e ancor più cruciali. Organizzare un evento sicuro

per le Regioni ospitanti, ma la sfida sarà anche quella di assicurare che questo stimolo sia distribuito equamente. A noi le sfide piacciono, sappiamo coglierle, sappiamo trasformarle in opportunità e sappiamo anche vincerle. Il cammino per l'organizzazione è cominciato un anno e mezzo fa, con il nostro Governo, perché ai Governi precedenti non importava, nonostante l'occasione speciale per l'Italia, malgrado avessimo preso un impegno e il fallimento dell'organizzazione avrebbe rappresentato un danno incalcolabile alla nostra immagine. D'altronde, era già capitato: ricordiamo tutti l'autoesclusione di Torino e la rinuncia alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, che invece si terranno quest'estate a Parigi. Fu come ammettere che non eravamo all'altezza non solo della realizzazione di grandi eventi nella capitale, ma anche di avere quella capacità di controllo per evitare che appalti finissero in mani sbagliate, nelle mani della criminalità organizzata (lo dissero loro, non certo noi). Insomma, invece di combattere la corruzione, il partito degli immacolati ha preferito alzare bandiera bianca per manifesta incapacità. Ancora una volta, la sinistra è capace di prevedere il futuro e chissà come mai sulle Olimpiadi prevede catastrofi e cataclismi, anche con un pizzico di sadismo misto a speranza che tutto vada storto. Mi chiedo davvero come si faccia ad essere così autolesionisti, raggiungendo un livello di anti-italianità davvero masochista. Questa è la differenza abissale tra noi e voi. Noi restiamo convinti che una buona riuscita dei Giochi convenga a tutti, al nostro Paese, alla nostra bandiera, perché saranno un biglietto da visita italiano all'estero. Voi, invece, sperate che queste Olimpiadi si trasformino in una macchia sulla reputazione, ma badate bene: a farne le spese sarebbe la reputazione di una Nazione, non di uno schieramento politico. *(Applausi)*. Questi Giochi - piaccia o non piaccia - sono figli di tutti noi. Non c'è proprio nulla da fare, voi - come avete già dimostrato - siete l'Italia dei no: no a nuove infrastrutture, no al Mose, no ai termovalorizzatori, no alle Olimpiadi a Roma, no all'alta velocità, no al Ponte sullo Stretto, no al TAP. Noi, invece - come abbiamo sempre dimostrato - siamo l'Italia dei sì: sì all'ammodernamento e alla creazione di ponti, strade, ferrovie per mettere fine ai viaggi della speranza dal Nord al Sud e perché il Paese abbia finalmente una dimensione europea; sì ad ogni strumento che permetta all'Italia l'approvvigionamento delle fonti energetiche di cui abbiamo così bisogno, con costi contenuti e benefici per tutti i cittadini. È la visione che vi manca perché, se fosse per voi, l'Italia tornerebbe indietro all'età della pietra; ma, poiché finalmente al Governo c'è il centrodestra, il nostro sguardo è proiettato verso il futuro le Olimpiadi rappresentano un modo per mostrare al mondo il progresso, l'eccellenza, la capacità organizzativa di un popolo che non merita di essere condannato alla mediocrità e all'immobilismo, ma stimolato ed esaltato per i suoi straordinari valori umani e professionali. Visto che parliamo di sport, userò termini sportivi. Ci sono due modi per affrontare una competizione: ritirarsi, cioè arrendersi e lasciare sulle spalle di chi ci ha preceduto tutta la responsabilità del fallimento, oppure mettersi ai blocchi di partenza e dimostrare di arrivare al traguardo e magari arrivarci per primi. Conosciamo i problemi e le difficoltà di un percorso cominciato nel 2019, quando fu assegnata all'Italia l'organizzazione dei Giochi, ma conosciamo anche la grande occasione che abbiamo davanti. Avremo modo di mostrare al mondo l'eccellenza del nostro sistema industriale, ingegneristico, manifatturiero, delle nostre materie prime, dei nostri prodotti. Abbiamo gli occhi di tutto il mondo puntati addosso, perché queste Olimpiadi saranno viste in TV da tre miliardi di spettatori e sapremo dimostrare il nostro valore, sapremo arrivare dove nessuno credeva possibile. Milano Cortina 2026 sarà un catalizzatore per investimenti in infrastrutture, trasporti e servizi, che avranno un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini ben oltre la conclusione dell'evento. Ci saranno benefici per il turismo, che aumenterà in modo esponenziale; le opere pubbliche, naturalmente, non saranno finalizzate soltanto ai Giochi; la nuova rete stradale e ferroviaria rappresenterà l'eredità che le Olimpiadi lasceranno al nostro Paese. È proprio su queste opere che interviene il decreto-legge che ci apprestiamo a votare oggi, sulla *governance* e sulle competenze dei lavori. Insomma, la macchina organizzativa marcerà a pieno regime. Non stiamo lasciando nulla al caso, pur fra mille contrasti e ostilità. A tal proposito, desidero ricordare che due settimane fa il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, ha ricevuto una lettera con minacce di morte: se vai avanti con la pista da bob, ti facciamo fuori. Questa lettera ha ottenuto l'effetto contrario, perché il sindaco Lorenzi ha annunciato l'intenzione di lavorare con ancora più determinazione. Quindi bravo sindaco, avanti così! il Governo e la maggioranza andranno avanti così, faranno ogni intervento possibile per rimuovere altri eventuali ostacoli, per agevolare la conclusione dei lavori, per poter tagliare i nastri di tutte le strutture dei Giochi olimpici anche prima delle scadenze previste. già detto, non ci fanno paura le sfide, alle quali tra l'altro siamo abituati, così come siamo abituati a lavorare, anche se circondati da chi vuole ostacolare noi e il nostro lavoro, che si tratti di Olimpiadi, di politica interna, di politica estera, di economia. Noi abbiamo l'ambizione di diventare un esempio di operatività, di efficienza e di capacità per tutti gli altri Paesi, non solo quelli europei. Tutti dovremmo fare il tifo per una buona riuscita delle Olimpiadi, perché decine di migliaia di nostri giovani sportivi le vedono come un traguardo, come un sogno. Milioni di cittadini aspettano l'accensione della fiamma olimpica con grande emozione e seguono con trasporto e passione ogni competizione. È questa la magia dei Giochi e noi questa magia la trasformeremo in realtà. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Faccio presente che l'assegnazione delle Olimpiadi invernali è avvenuta sotto il Governo Conte, con il MoVimento 5 Stelle, non è questo. Il fatto è che gli obiettivi sono condivisi, nel senso che tutti approviamo questo intervento, ma le modalità e le tempistiche, viceversa, non ci convincono. Io ho ancora chiara nella mente l'immagine del sindaco di Milano, Beppe Sala, al momento dell'assegnazione delle Olimpiadi. La sua esultanza

e quella ambientale, anche nell'ottica della cosiddetta *legacy* (non avevo mai sentito usare tanti termini anglofoni quanto con questo Governo, che aveva esordito col dire che non si sarebbero dovuti usare).

sfida interconnessa dei trasferimenti, dei trasporti. Pertanto, il popolo delle Olimpiadi, gli atleti con i loro *team*, i giornalisti, gli organizzatori, le autorità dovranno spostarsi in questo quadrilatero,

Quale occasione migliore da cogliere se non questo evento sportivo per lasciare sul territorio l'eredità di un miglioramento dei servizi di trasporto? È una cosa che purtroppo - ahimè - non accadrà,

neanche un euro alla realizzazione di nuove tratte ferroviarie. Quello che viene speso per i servizi ferroviari concerne l'eliminazione dei passaggi a livello.

Pochi chilometri da superare e si sarebbe potuta raggiungere Cortina da Venezia e da Belluno esclusivamente con il treno. Stessa cosa dall'altra parte in Lombardia: tra Tirano e Bormio manca un pezzettino, ma non se ne è fatto nulla. saremo costretti a raggiungere le località con mezzi di trasporto su gomma (quindi su strada), congestionando il traffico e aumentando l'inquinamento. Attenzione, perché siamo in un territorio che è sotto procedura di infrazione - solo qualche giorno fa ne è stata aperta un'altra - per superamento delle soglie di inquinamento. Sappiamo benissimo che la circolazione dei veicoli incide notevolmente sulle sostanze inquinanti emesse. Quindi, cogliendo l'opportunità delle Olimpiadi, si sarebbe potuto rispondere anche a questa esigenza: togliere veicoli inquinanti dalle strade e implementare il servizio di trasporto su ferro. *(Applausi)*. Questo era un investimento utile da fare. un altro esempio: la pista da bob di Cortina è stata individuata come una priorità, come uno di quegli interventi indifferibili e urgenti da raggiungere costi quel che costi, costerà un sacco di soldi. La programmazione è quella di realizzare un'opera nel giro di poco più di quasi due anni, lavorando giorno e notte, sette giorni su sette, pur di realizzare l'obiettivo. Queste sono scelte politiche; l'ordine delle priorità lo dà la politica. Non sarebbe stato meglio investire cotanta energia nella realizzazione dei tratti ferroviari mancanti, che avrebbero risposto alla duplice esigenza di trasferire il popolo delle Olimpiadi e successivamente, come eredità,

utili. Tornando alla pista da bob, la senatrice Ronzulli parlava dell'immagine dell'Italia, dell'efficienza e della capacità organizzativa.

Eugenio Monti delle Olimpiadi del 1956, è stato dismesso dal Comune di Cortina perché non era sostenibile economicamente. Banalmente uscivano molti più soldi di quanti ne entrassero, quindi nel 2008 l'hanno chiusa. Stessa sorte ha subito la pista da bob di Cesana, in occasione delle Olimpiadi del 2006 a Torino. Allora c'è qualcosa che non va, perché *repetita non iuvant*. non c'è due senza tre - faremo la terza pista inutile, perché gli atleti che si dedicano a questo sforzo sono veramente pochissimi, perché vanno ad allenarsi già da tempo altrove e continueranno ad allenarsi altrove. manutenzione e una gestione costosissime che il Comune non si può permettere, quindi nel giro di qualche anno tornerà ad essere un rudere, non senza prima aver abbattuto un bosco di 500 larici secolari e devastato un territorio che del paesaggio fa il suo vanto. Ricordo che il ministro Giorgetti ha manifestato qualche perplessità. Le sfide si colgono, ma previa valutazione, perché buttarsi in un baratro non è una sfida, ma un atto demenziale. Ormai il bosco è stato abbattuto, con violoncellista di sottofondo e con pianti dei residenti. Vedremo che cosa accadrà. Tra l'altro, se non si arriverà per tempo alla consegna di quest'opera, il che non è per niente improbabile, dovremo comunque rivolgerci all'estero. Quindi avremo speso il doppio dei soldi e ottenuto praticamente un risultato inutile. queste Olimpiadi creeranno posti di lavoro. Apro una parentesi divertente: chi lavora per la pista di Cortina? Vi lavorano 90 operai norvegesi, perché gli italiani non si sognano di lavorare a quelle temperature. Quindi, i posti di lavoro della pista di Cortina andranno ai norvegesi e gli italiani rimarranno a casa. a casa. Per quanto riguarda le tratte ferroviarie, tra le opere indifferibili e urgenti non è stato preso in considerazione, per esempio, il collegamento dell'aeroporto Orio al Serio alla città di Bergamo: il che significa di nuovo che dovremo usare il trasporto su gomma, andando ad appesantire ed aumentare l'inquinamento. Questa era un'opera prioritaria e indifferibile, come lo erano le altre due di collegamento, ma sono state accantonate. È stato dato l'appalto ad ANAS per la costruzione in velocità delle strade, perché questo Governo ha una caratteristica: si muove in emergenza, non si riesce neanche a capire di che cosa si sta parlando. Adesso ANAS ha l'appalto delle strade e dovrà fare tutto in velocità, superando tante attenzioni che, viceversa, sarebbero dovute nel momento in cui si va ad incidere su un territorio che è già al collasso a livello di viabilità su strada e di impermeabilizzazione del suolo. Avevo chiesto negli suolo. Avevo chiesto negli emendamenti che venisse redatto un bilancio economico, ecologico ed ecosistemico, in modo da valutare la situazione che si creerà. L'ideale era farlo in via preventiva; non pretendo questo, ma quantomeno a fine delle opere, in modo da capire che cosa rimane sul territorio, quella famosa eredità. Avevamo chiesto in estremo subordine, visto che non vengono considerate le nostre opzioni, di creare almeno un piano e una programmazione per l'interconnessione del trasporto pubblico, per evitare che si creino disagi e intoppi. Ma non è stato fatto nulla: la flotta del mezzo di trasporto pubblico, in modo che fosse a basso impatto ambientale. Niente di questo è stato fatto. Fondamentalmente, sul nostro territorio rimarrà un'eredità.

il decreto-legge su cui oggi siamo chiamati a esprimerci ha l'obiettivo di garantire che le opere infrastrutturali di trasporto, indispensabili per poter ospitare i Giochi olimpici, siano completate con certezza e nei tempi necessari. È chiaro infatti che non solo lo svolgimento delle Olimpiadi, ma anche il loro successo e la buona riuscita non possono che passare attraverso un'adeguata rete di infrastrutture e anche di trasporti, così da rendere facilmente raggiungibili e fruibili per chiunque le località in cui si svolgeranno le gare. Per farlo abbiamo ritenuto che fosse fondamentale e non più procrastinabile agire innanzitutto sulla *governance* della Simico, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, prevedendo una sua ristrutturazione, ma non perché - come qualcuno ha ipotizzato poc'anzi - volessimo mettere "le mani in pasta" - credo che non sia il modo di fare politica di questo Governo *(Applausi)* e lo sta dimostrando con le azioni ma perché, appunto, per via dei ritardi sui quali tutti ci troviamo d'accordo, erano necessarie una ristrutturazione della *governance* e una revisione delle attribuzioni commissariali. Questo per assicurare simultaneamente una gestione efficiente, trasparente e celere dei processi decisionali, da da un lato, e una corretta allocazione delle risorse pubbliche, dall'altro. Quindi, l'approvazione di questo provvedimento rappresenta un passo fondamentale per massimizzare i benefici derivanti all'intero Paese dall'organizzazione dell'evento. Voglio sottolineare cosa vuol dire e che significato hanno per l'Italia nel suo complesso i Giochi olimpici e paralimpici invernali sul territorio. Questa grandiosa manifestazione, che richiama atleti appassionati da tutto il mondo, non riguarda ovviamente solo la Lombardia o il Veneto, ma rappresenta un'opportunità straordinaria

per ospitare le Olimpiadi, a differenza di quanto accaduto a Roma qualche anno fa, quando la miopia di una certa parte politica ci ha fatto perdere una irripetibile opportunità. Quindi, dal punto di vista economico, è chiaro che l'organizzazione dei Giochi olimpici rappresenta un impulso significativo per il PIL italiano. Si genera infatti, già nell'immediato, un flusso di attività che coinvolge numerosi settori, dall'edilizia alla logistica, dal turismo all'intrattenimento e via dicendo, che comporta

dal punto di vista del prestigio internazionale e dell'immagine che ne viene trasmessa, si tratta di un'opportunità unica per l'Italia di mostrare al mondo la ricchezza culturale e la bellezza del proprio territorio, nonché anche - perché no? - le proprie capacità organizzative. L'attenzione mediatica mondiale, riservata in particolare proprio agli eventi sportivi, offre in questa occasione una vetrina senza pari per promuovere i valori italiani anche di inclusione, di solidarietà e passione per lo sport, diventando anche un modello da poter replicare poi

nella realizzazione delle opere infrastrutturali con l'attenzione verso le esigenze delle comunità coinvolte e il valore, appunto, che tale evento assume per tutti noi. Nella mia veste di Capogruppo della Lega in Commissione trasporti e in linea con l'azione promossa dal ministro Salvini, non posso non rimarcare

come sappiamo - il tempestivo completamento delle opere previste per poter ospitare, come richiede un intervento internazionale di tale portata, infrastrutture di alta qualità assieme a una gestione impeccabile e a una pianificazione curata in ogni dettaglio, perché dobbiamo offrire un contesto adeguato e sicuro per accogliere atleti e spettatori di tutto il mondo. A questo fine, gli emendamenti approvati dall'8a Commissione si sono concentrati in particolare sul potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, con la designazione di RFI come soggetto responsabile.

passaggi a livello della SS 38, che - come sappiamo - sono purtroppo fonte di enormi rischi, troppo spesso sfociati in tragedia anche di recente. Quindi garantiamo, attraverso questa previsione, la sicurezza e la fluidità del trasporto su strada durante l'evento. È degna di nota anche l'assegnazione alla società Ferrovie Nord della responsabilità per il collegamento tra il Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa e la rete ferroviaria nazionale; intervento che rappresenta un passo di estrema importanza nel preparare l'infrastruttura per i Giochi. Questo collegamento infatti non solo favorirà lo spostamento agevole di persone e risorse, ma contribuirà anche in modo significativo al successo logistico complessivo dei Giochi. RFI, poi, avrà un ruolo chiave, per noi importantissimo, nell'attuazione di specifici interventi su ulteriori aspetti riguardanti le esigenze degli atleti e delle persone con disabilità. Questo punto rappresenta una grandissima conquista di civiltà. Voglio ricordare oggi l'incessante impegno che viene soprattutto dal mio partito nei confronti della disabilità, con un Ministero dedicato, oggi mirabilmente ricoperto dal ministro Locatelli e in precedenza dalla ministra Stefani *(Applausi),* per promuovere l'inclusione e rimuovere le barriere architettoniche, di cui ancora oggi il nostro Paese è purtroppo disseminato, che impediscono la piena partecipazione alla vita quotidiana delle persone con disabilità. La Lega, invece, dimostra un'attenzione continua e concreta nel promuovere l'accessibilità e l'inclusione di tutti mediante interventi infrastrutturali mirati, ma anche adoperandosi in uno sforzo continuo per sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni sui diritti e i bisogni delle persone con disabilità, promuovendo promuovendo politiche e progetti mirati a migliorarne la qualità della vita. È in questo solco, nel contesto dei Giochi olimpici e paraolimpici, che l'impegno per l'inclusione si materializza nella progettazione e realizzazione di infrastrutture che siano conformi ai più elevati *standard* di accessibilità. Ciò implica non solo la realizzazione di strutture sportive e di accoglienza idonee, ma anche l'ideazione di soluzioni innovative per superare le barriere in generale e facilitare anche l'utilizzo degli spazi. Questo perché i diritti delle persone con disabilità devono essere sempre garantiti, ma a maggior ragione in occasione di

piena funzionalità e fruibilità, nonché il regolare svolgimento dell'evento. Infine, abbiamo rivolto la nostra attenzione, con l'ultimo emendamento approvato in Aula, anche allo stato dei luoghi, prevedendo che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali provveda all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per contrastare il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo al territorio del Comune di Cortina. Tale aggiornamento è senz'altro strategico nella gestione ottimale del territorio in vista

un piccolo particolare, cioè il fatto che le *mascotte* olimpiche e paraolimpiche, rappresentate dai due tenerissimi ermellini, Tina e Milo, sono state ispirate dal talento di alcuni giovani della mia terra. Tina e Milo, infatti,

Io ho incontrato i ragazzi e li voglio qui ricordare, anche per il significato che le *mascotte* hanno, dal momento che incarnano i valori di inclusione e di rispetto per le diversità e di amore per la natura, cioè lo spirito più autentico dei Giochi olimpici e paraolimpici, che si fonda su una competizione reale, volontà di superare le sfide e sul potere unificante dello sport, che appunto unisce le persone di ogni genere e provenienza verso un unico obiettivo. Per tutto questo, quindi, è essenziale che questo decreto-legge in esame sia approvato senza ulteriori indugi. valori passano, infatti, anche per il completamento tempestivo delle infrastrutture necessarie a consentire lo svolgimento dei Giochi nella migliore maniera possibile. A conferma del nostro impegno costante e del lavoro instancabile che stiamo portando avanti in questa direzione, esprimo, a nome del Gruppo Lega, il nostro voto, che non può essere

il decreto che stiamo discutendo è indubbiamente cruciale per consentire il completamento, nei tempi previsti, delle opere legate all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali. Lo hanno detto tanti colleghi: quello di cui stiamo discutendo è un evento di grande portata, di livello internazionale; un evento molto impegnativo, anche dal punto di vista economico. La spesa è pari a 3,6 miliardi, tra fondi pubblici e fondi privati. Noi saremo in vetrina nei momenti in cui si svolgeranno le Olimpiadi. Ne va della nostra immagine. Le Olimpiadi sono una grande opportunità di crescita economica, di creazione di lavoro e di sviluppo infrastrutturale per i territori interessati.

che riguarda tutti. Mi rivolgo, attraverso lei, Presidente, alla senatrice Ronzulli. Qui non c'è un noi e un voi, chi è contro e chi a favore: qui facciamo tutti il tifo per l'Italia. Facciamo tutti il tifo per la realizzazione di queste opere e nessuno può chiamarsi fuori, perché - come è stato ricordato - le Olimpiadi sono state assegnate con il Governo Conte, si sono susseguiti i Governi di ogni colore politico; le Regioni Lombardia e Veneto sono da tanti anni governate dalla destra e molti enti locali dal centrosinistra. Tutti siamo corresponsabili e ci dobbiamo sentire tali per il successo di questo grande evento. Presidente, noi siamo preoccupati, siamo molto preoccupati per i tempi di realizzazione delle opere e per la modalità di realizzazione delle infrastrutture. Suggerisco ai colleghi della maggioranza di lasciar perdere la retorica e la propaganda perché servono a poco. Serve a poco la retorica e serve ancora meno attaccare le forze che si collocano all'opposizione, come se noi fossimo i disfattisti che tifano contro. Non è così e cercherò di argomentarlo. Qui è in gioco l'immagine del Paese. Abbiamo ragione però di essere preoccupati non per disfattismo, ma per quello che abbiamo letto da ultimo nelle considerazioni della Corte dei conti del Veneto non di dieci anni fa, ma di tre settimane fa. La Corte dei conti del Veneto ha evidenziato il ritardo nelle attività rimesse alla Simico SpA e infatti il provvedimento decide il subentro di ANAS. La Simico infatti non ce la faceva palesemente a svolgere i compiti che le erano stati affidati. La Corte ha evidenziato altresì il ritardo di due infrastrutture cruciali, come la variante di Cortina e quella di Longarone, che valgono 800 milioni di euro da sole di investimenti; le spese della Fondazione Milano Cortina e, da ultimo, non ultima in ordine di importanza, la patetica telenovela della nuova pista da bob di Cortina che, da sola, la dice lunga sulle vicissitudini di questi Giochi olimpici. Dico con grande nettezza che, come senatori e senatrici del Partito Democratico, noi ci sentiamo impegnati, sentiamo come un nostro dovere collaborare per il successo di questo evento. Ma sentiamo altrettanto la responsabilità e il dovere di batterci perché le opere infrastrutturali, centinaia di milioni di opere infrastrutturali, siano realizzate nel pieno rispetto di alcuni principi: la trasparenza, l'efficienza la sostenibilità. Sono in gioco tanti soldi pubblici e un'eredità positiva che dobbiamo lasciare a quei territori e alle generazioni future. Questa discussione rappresenta allora un'occasione per fare il punto su quello che ha funzionato e soprattutto su quello che non sta funzionando e che va corretto. Il provvedimento in esame contiene una serie di scelte condivisibili, come abbiamo detto nel corso della discussione in Commissione e negli interventi che si sono succeduti in Assemblea. Lo ribadiamo anche in questa dichiarazione di voto, ma non possiamo non evidenziare alcune preoccupazioni che ci spingono in una posizione di cautela. Siamo preoccupati della trasparenza nelle procedure di affidamento delle opere e non ci basta quanto è previsto da questo decreto-legge. Siamo preoccupati per l'impatto ambientale di questi progetti infrastrutturali, perché l'accelerazione è indispensabile, altrimenti non arriviamo in tempo. Attenzione però all'impatto ambientale. poi il tema molto importante della reale distribuzione dei benefici economici tra le comunità locali, perché le modifiche alla *governance* della società Infrastrutture e l'accentramento di alcune funzioni rischiano di escludere dal processo decisionale le realtà locali, che invece devono essere coinvolte nei processi per la buona riuscita di questo straordinario progetto. Queste preoccupazioni ci hanno portati a presentare, con spirito costruttivo, una serie di proposte emendative e a chiedere dei chiarimenti nel corso della discussione. Alcune delle nostre proposte sono state accolte - ne diamo atto al Governo e alla maggioranza - come ad esempio quella sul tema dell'individuazione di Ferrovie Nord quale soggetto attuatore o come l'emendamento che consente agli enti territoriali interessati dai Giochi di concorrere a finanziare e a svolgere attività inerenti. Abbiamo presentato un emendamento per assegnare agli enti territoriali competenti le opere di carattere permanente, che è stato trasformato in un ordine del giorno accolto dal Governo. Altre proposte - ahinoi - sono state respinte. Nel complesso - lo voglio ribadire - continueremo a porci con spirito collaborativo e costruttivo nei confronti di questa iniziativa. iniziativa. In conclusione, signor Presidente, ribadisco i punti salienti della posizione del Partito Democratico, che ci hanno guidato nella discussione in Commissione e che continueranno a guidarci nei meno di due anni che mancano per l'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici. È un evento di portata strategica per il Paese, di grande portata economica, sociale e infrastrutturale. È una vetrina per il nostro Paese, e dobbiamo esserne consapevoli. dobbiamo esserne consapevoli. Dobbiamo mettere in condizione innanzitutto i territori interessati di cogliere tutte le opportunità offerte dai quasi quattro miliardi di euro di investimenti e da ciò che verrà generato dai Giochi in termini turistici e di attività di quei territori, ma chiediamo al Governo di fare di più in relazione alle preoccupazioni che ho esposto in questo intervento. Noi ci asterremo nel corso della votazione, signor Presidente, innanzitutto per queste motivazioni. Facciamo il tifo per la riuscita e per il successo di questo evento. Siamo disponibili a collaborare con spirito costruttivo, con le proposte che abbiamo presentato e con quelle che continueremo ad avanzare, ma chiediamo al Governo un approccio più equilibrato, che consideri fino in fondo tutte le variabili che sono in gioco a livello nazionale e a livello territoriale. È per questo che il Gruppo Partito Democratico si asterrà dal

festeggiammo la designazione di Cortina e Milano - uso il rigoroso ordine alfabetico, quindi non me ne vogliano i colleghi lombardi - quale sede delle Olimpiadi. di un grande lavoro che ha messo insieme sostanzialmente tutto l'arco alpino. Ricordo che per farsi assegnare le Olimpiadi fu redatto un *dossier*, all'interno del quale c'erano le opere che ci saremmo impegnati a

sottolineo l'arco alpino perché queste, nonostante siano le Olimpiadi di Cortina e di Milano, hanno una diffusione ampia, quasi fosse un un'area vasta - tornerò sulla questione dell'area vasta, perché non uso questo termine a caso perché anche le Province vicine, come la Provincia di Belluno in questo caso, dove ha sede Cortina, saranno sede di attività sportive, e lo dico con orgoglio. Lo dico con orgoglio, perché sullo sport e su una questione così importante come le Olimpiadi non possiamo avere confini geografici che ci dividono; anzi, anzi, non possiamo avere confini ideologici che ci dividono. Dico questo a beneficio di chi è intervenuto poc'anzi, in maniera un po' polemica, circa il fatto che il Governo faccia o non faccia propaganda. In realtà, quale rappresentante del Gruppo più numeroso di quest'Assemblea, faccio appello allo spirito olimpico e dico una cosa che può sembrare banale, ma noi abbiamo fatto una grande fatica. Fratelli d'Italia era all'opposizione nel 2019, ma ha sempre creduto fortemente in questi Giochi olimpici. Lo ha fatto, appunto, dall'opposizione, a testimoniare che non abbiamo bisogno di ribadire che siamo a favore dell'Italia e che tifiamo per l'Italia. Lo facciamo con gli atti formali, con le presenze in Parlamento e anche con i nostri voti. Lo dico perché queste Olimpiadi hanno messo insieme la potenza commerciale e politica di Milano e della Lombardia con il grande blasone, il nome, la storia, la bellezza di Cortina, la perla delle Dolomiti. Lasciatemelo dire: io vivo a pochi chilometri da Cortina e sono orgoglioso che si possa replicare quello che si fece nel 1956. Se oggi Cortina è riconosciuta universalmente nel mondo non solo come la perla delle Dolomiti, ma anche come un *brand,* lo si deve al fatto che nel 1956 noi facemmo una grandissima bella figura e tutto il mondo, ancora oggi, anche e soprattutto negli Stati Uniti, ci riconosce la straordinaria capacità di vendere l'italianità, anche in montagna. Da Da quella data però, dal 19 giugno - come ha detto il collega Rosa, che ha seguito i lavori in 8a Commissione

ma anche supportato in queste Aule da tutte le forze politiche. È per questo che ora qualche distinguo, forse anche un po' ideologico, ci fa pensare che sia solo strumentale e non sostanziale. *(Applausi)*. se qualcuno può pensare che qualcuno faccia un distinguo di questo tipo: lo fa perché gli atti fino al 26 settembre 2022 vedevano tutte le forze politiche che componevano la maggioranza assolutamente coese.

ad ANAS in questo caso - un quadro che prevede che si possano fare affidamenti molto più veloci, sempre nel rispetto delle normative - lo dico da sindaco, non da senatore in questo caso

nel corso di questi anni possa vedere realizzare il frutto del proprio lavoro. È questo l'appello che faccio: non dividiamoci, vi prego, su questa tematica, perché altrimenti daremmo

non solo una ricaduta lavorativa, né soltanto una ricaduta di immagine, ma anche l'unica speranza per invertire una tendenza, quella dello spopolamento, che in certe aree interne, compresa la mia, ha preso il sopravvento da tempo. Il mio è un appello accorato. Potevamo fare di più? Si poteva fare di più? Sì, si può sempre fare di più e questo decreto-legge ne è la dimostrazione. Però dico alla senatrice Sironi, che citava la linea ferroviaria Calalzo-Cortina - e glielo dico non da senatore della Repubblica, ma da sindaco di Calalzo io avrei chiaramente gradito e voluto che ci fosse la ferrovia a Cortina-Calalzo, che tra l'altro una volta esisteva, ma su di essa abbiamo costruito un'altra un'altra infrastruttura, tanto decantata e che ho sentito nominare anche durante la discussione generale, cioè una pista ciclabile. Allora delle due l'una: manteniamo la pista ciclabile più bella del mondo, quella che da Calalzo va a Lienz, oppure ci facciamo la ferrovia? Se avessimo avuto tempo e risorse per fare anche la ferrovia, credo che non avreste trovato nessuno contrario. Ma se aveste chiesto a qualsiasi cittadino della provincia di Belluno

citato non solo la circonvallazione di Cortina, ma anche quella di Longarone, che funge da tappo non solo per i turisti al ritorno, ma anche per i tanti residenti - se avessimo messo questi elementi sulla bilancia; se avessimo fatto un qualsiasi *referendum* così caro a tante forze forze politiche, i cittadini non avrebbero avuto alcun dubbio: tutti avrebbero voluto una viabilità che funziona. Quando mi sento dire - senatrice Aurora Floridia, lei sa quanto io le voglia bene - che 3 miliardi dedicati alle strade non sono un beneficio che rimarrà alle comunità locali, le dico che le strade e le infrastrutture da sempre rappresentano uno

per l'appello allo spirito olimpico che sono sicuro che in quest'Aula alberghi, dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

colleghi, quando il nostro capo politico Giuseppe Conte ottenne per l'Italia oltre 200 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, chiarì che circa la metà delle risorse era destinata per il Sud Italia. Del resto, questo importo così imponente fu erogato adottando tre parametri: il PIL *pro capite*, la popolazione residente e il tasso di disoccupazione, che avevano proprio l'obiettivo di mettere in moto la locomotiva meridionale. Ma mi chiedo: come stiamo impegnando questi fondi? Male, anzi direi malissimo e la cosa più grave è che la cabina di regia sul PNRR è detenuta da un Ministro meridionale. Devo ammettere che sta davvero mettendo tutto il suo impegno per sprecare questa occasione di sviluppo per la nostra terra. Onorevoli colleghi, ricordo che la maggior parte di tali fondi dovrà essere utilizzata entro il 2026, pena la restituzione delle risorse alla Comunità europea. Ebbene, qual è l'importo utilizzato fino ad oggi? Briciole. Basti pensare che, secondo un'inchiesta pubblicata negli ultimi giorni da «Il Sole 24 Ore», nella relazione semestrale presentata dal Governo sulla spesa effettiva del PNRR, la spesa effettiva ad oggi è di appena di 45,6 miliardi di euro. Tuttavia, oltre il danno c'è la beffa, o meglio, l'inganno. Sempre secondo il quotidiano economico «Il Sole 24 Ore», questo importo include 26,7 miliardi di euro utilizzati per pagare i crediti di imposta dei superbonus, per Industria 4.0 e per incentivi a ricerca e sviluppo: somma che non riguarda alcun nuovo investimento, né alcuna opera pubblica per cui il PNRR era stato pensato. Sapete che significa? La spesa reale complessiva 2021-2023 si è fermata ad appena 18,9 miliardi di euro, cioè il nostro Paese ha speso ad oggi soltanto l'11 per cento dei fondi e ora toccherà spenderne l'89 per 151 miliardi entro il 2026. La cosa grave è che il ministro Fitto non ha negato questo imbroglio contabile, ma - peggio puntato il dito contro gli enti pubblici e la piattaforma ReGis, che avrebbe - a suo dire - falsato le cifre degli investimenti in opere pubbliche, ben più consistenti. anche se fosse vera la tesi del ministro Fitto, perché appena insediatosi non è intervenuto per correggere le criticità di questa piattaforma? I dubbi e le perplessità sono tante, anzi tantissime, motivo per cui ho depositato un'interrogazione parlamentare con cui ho invitato l'esponente pugliese a riferire non solo alla senatrice Aloisio, non al MoVimento 5 Stelle, ma a 60 milioni di italiani.

onorevoli colleghi, voglio esprimere profonda preoccupazione per le gravi condizioni che stanno affrontando i cittadini di Cuba nelle ultime ore. L'Isola sta vivendo la più severa crisi alimentare ed energetica dalla rivoluzione comunista del 1959, con conseguenze disastrose per tutta la popolazione. A fronte di questo, è in atto una vera e propria *escalation* di proteste da parte del popolo contro il regime di Raul Castro e Diaz-Canel; proteste iniziate venerdì scorso a Santiago de Cuba e rapidamente diffuse in numerose città dell'Isola e già sotto la scure nera della repressione militare, come già avvenuto con le rivolte dell'11 luglio 2021. Quelle repressioni ci consegnarono più di 1.200 prigionieri politici, e cioè persone mandate in galera solo perché non era consentito loro di esprimere il dissenso contro la dittatura comunista. Tra quei prigionieri ci sono ancora più di 100 bambini. Oggi gli abitanti di Cuba, già oppressi da una povertà dilagante, da un'inflazione incontrollabile, stanno affrontando una situazione umanitaria critica, con la mancanza di beni di prima necessità come il latte e il pane, i cui prezzi sono diventati proibitivi. A ciò si aggiunge l'inaccettabile aumento del 500 per cento del prezzo della benzina, decisione che ha ulteriormente peggiorato la loro vita quotidiana. Tomoya Obokata, relatore speciale per le forme di schiavitù contemporanee, ha indirizzato alla rappresentanza dell'Avana un documento per attirare l'attenzione sui modelli persistenti a Cuba, che ricordano il lavoro forzato, come da definizione dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Inoltre, la decisione del Governo di interrompere le comunicazioni e l'accesso a Internet rappresenta un chiaro e inequivocabile tentativo di isolare i ribelli e impedire al mondo esterno di conoscere la gravità della situazione. Noi abbiamo notizie che arrivano dagli esuli in Italia da parte dei familiari che cercano di oltrepassare i vincoli delle reti VPN e di riprendere quanto sta accadendo, anche tenendo conto del razionamento dell'energia elettrica che da due anni a questa parte sta diventando più esiguo. L'Osservatorio cubano per i diritti umani avverte che le proteste di massa delle ultime ore in diverse città cubane finiranno in tragedia, se non si avvieranno immediatamente i cambiamenti politici, economici e sociali. Cuba non è l'isola felice e patinata descritta dalle cartoline turistiche. La realtà consiste in un popolo costretto a condizioni di vita disperate, senza più alcuna assistenza, senza cibo, senza elettricità. Questo nonostante gli ingenti aiuti umanitari forniti per decenni dagli Stati occidentali. Di contro, nella piramide della società cubana, troviamo un regime castrista che impiega fiumi di denaro per il proprio personale tornaconto e per il rafforzamento dell'apparato di repressione, nutrendo il proprio consenso con arresti e processi sommari, così come ben argomentato in più rapporti di organizzazioni internazionali quali Amnesty International. Infine, lo scorso autunno è emerso anche da alcune coraggiose testimonianze di giovani cubani il loro essere stati illusi di ricevere un passaporto e la cittadinanza russi per trovare un lavoro lì, per poi essere privati dei documenti e mandati con l'inganno a combattere al fronte in prima linea contro l'esercito ucraino. Questo a dimostrare quanto sia ancora forte e indipendente il rapporto tra il regime cubano e quello russo. Concludo esprimendo piena solidarietà a tutto il popolo cubano e auguro loro finalmente un futuro dignitoso e libero. *Patria y vida*.

che sarebbero state riscontrate nella scuola Iqbal Masih di Pioltello. Per intenderci, la scuola che avrebbe scelto un calendario scolastico votato all'unanimità e che, a quanto pare, presenta delle irregolarità. Vorremmo sapere quali sono, anche per evitare che altre scuole, eventualmente, possano incorrere nell'errore formale della formulazione del calendario scolastico. Quindi il Ministro dovrà venire qui a spiegarci, per aiutare anche le altre scuole ed eventualmente a correggersi sulle interpretazioni. Approfitto di di questi pochi minuti, perché oggi il Ministro alla fiera Didacta Italia ha parlato nuovamente della scuola di Pioltello, dando dati parziali e dicendo che è una scuola che ha risultati molto bassi per quanto riguarda l'Invalsi. Vorrei ricordare al Ministro che l'Invalsi elabora dati attraverso comparazioni e che bisognerebbe guardare qual è il criterio che è stato utilizzato, cioè l'indicatore ESCS che definisce lo *status* sociale, economico e culturale delle famiglie degli studenti. Quindi per Invalsi si devono comparare dati che appartengono, diciamo così, agli stessi bacini di questo indicatore. Il Ministro si è dimenticato di dirlo, perché se si comparano invece i i dati di questa scuola con tutte le altre scuole d'Italia che hanno lo stesso tipo di bacino e quindi di indicatore, siamo ben sopra la media perché, per esempio, i bambini ottengono più 23,3 in matematica, più 27,6 in inglese per l'ascolto, più 23,2 in inglese per la lettura e, sì, meno 0,1 punti per quanto riguarda le prove di di italiano, anche perché le prove di italiano Invalsi devono essere fatte da tutti gli studenti, anche dai cosiddetti NAI, cioè dai neoarrivati in Italia da meno di due anni, che quindi non sono alfabetizzati e che hanno un percorso di aiuto e di sostegno, ma che riescono comunque ad affrontare queste prove grazie a quella didattica che eventualmente funziona. L'ESCS di questa scuola è molto basso, perché si tratta di una scuola che è in un tessuto sociale che ha delle difficoltà e io vorrei, visto che il Ministro è andato a verificare questi dati, che adesso approfittasse di venire a Pioltello e di dare magari una mano ulteriore a quelle scuole che vivono in questa realtà per poterle aiutare.